Colleghi, come già sapete, nella giornata del 14 maggio la dottoressa Elisabetta Serafin è stata nominata...

di finire la frase che avete fatto l'applauso al nome, il che è più significativo di qualsiasi parola potessi pronunciare. Vuol dire che non c'è bisogno di ricordare quello che la dottoressa Serafin ha fatto per il Senato, per l'equilibrio, l'autorevolezza e la gentilezza con cui ha svolto questo delicatissimo incarico, che ricopre, se non mi sbaglio, dal febbraio del 2011 e che ha ritenuto di lasciare quando si avvicinava la scadenza, anche per rispondere a una prestigiosa chiamata quale quella di presidente della Saipem, una delle aziende italiane più importanti. Le ho chiesto io di essere oggi qui con noi, perché voi possiate salutarla con l'applauso che avete voluto già tributarle. Io l'ho conosciuta bene, come potete immaginare, ma come me l'hanno conosciuta diversi Presidenti che mi hanno preceduto,

capacità di unire alla competenza l'equilibrio, che è la cosa più difficile che ci possa essere e che si possa trovare. Anche il presidente Monti l'ha avuta come

i migliori auguri di buon lavoro di tutto il Senato, di tutti i senatori e mio personale.

ciascuno di noi che ha lavorato con la dottoressa Serafin possa manifestarle la grande riconoscenza per aver sempre lavorato a tutela dell'Amministrazione di cui ha fatto parte per tanto tempo, che credo porterà nel cuore anche in questo suo nuovo prestigiosissimo incarico.

In tutti i momenti anche complicati che abbiamo affrontato in questi anni, la dottoressa Serafin ha saputo sempre avere come unico obiettivo la tutela dell'Amministrazione e il bene pubblico nel

Signor Presidente, intanto vorrei ringraziarla per aver avuto questo gesto di cortesia nei confronti della dottoressa Serafin. esprimere, a nome personale e del Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe, il nostro ringraziamento, il nostro apprezzamento e i migliori auguri per l'importante incarico che è stata chiamata ad assolvere alla dottoressa Elisabetta Serafin, che vogliamo davvero ringraziare sia per il tratto con il quale ha voluto svolgere la sua importante attività e la sua significativa funzione, sia per il modo con cui ha assicurato un'assoluta e totale imparzialità e una capacità anche di supporto, non banale e non ordinaria, ai lavori che siamo chiamati ad assolvere e alle funzioni che il popolo ci ha assegnato. Più in generale, signor Presidente, credo che questo gesto corale di applauso vada certamente alla persona, ma lo vorrei anche interpretare come un gesto di apprezzamento nei confronti della funzione chi assolve tale funzione, unitamente alle altre funzioni di apicalità e di struttura, rappresenta un'intelaiatura essenziale, fondamentale, indispensabile per l'assolvimento e per l'equilibrio della nostra democrazia. In questi tempi in cui con troppa faciloneria si tende a generalizzare, un apprezzamento di questa natura credo abbia un valore doppio.

cui ha svolto il suo delicatissimo ruolo in questi anni. Credo sia importante per tutti, sia quando si è in maggioranza sia quando si è all'opposizione, sapere che nei funzionari del Senato, a cominciare dal suo vertice, il Segretario Generale, c'è chi dà tranquillità a tutti: si sa che le regole vengono osservate, le procedure attuate correttamente

Grazie Io sono neofita del Senato e quindi, purtroppo, ho potuto usufruire poco della capacità, della competenza, della grazia, del rispetto per le istituzioni che ha sempre apportato a quest'Aula la dottoressa Serafin, la cui fama, comunque, la precedeva anche nei tanti anni che io ho trascorso alla Camera. Devo dire che la saluto con un po' di magone, perché ho potuto apprezzarla tanto in questo anno e mezzo, da quando, appunto, sono qui al Senato. Anche a nome, ovviamente, del senatore Questore, che lei invece conosce da tantissimi anni, e a nome di tutto il mio Gruppo, le faccio i miei migliori auguri. È una È una persona che, appunto, ho imparato ad apprezzare. Credo che le sue doti straordinarie, anche di prima donna assurta ad un ruolo così importante all'interno delle istituzioni, l'accompagneranno anche, ovviamente, in questa sua nuova professionalità, in questa sua nuova mansione. È lei che ha aperto il varco - come

Signor Presidente, da parte nostra, come Lega, penso non basterebbe neanche un intervento di venti minuti, come consentito dal Regolamento ai Capigruppo, per poter esprimere tutta la nostra riconoscenza nei confronti della dottoressa Serafin

anche con questa sensibilità particolare, per far sì che tutte le strutture, tutti i funzionari del Senato, si trovassero a loro agio. Poi, tutte le strutture hanno sempre dei problemi, ed è normale che sia così, ma bisogna veramente riconoscere un grande merito a tutto il lavoro che

anche la postura che un Capogruppo e un senatore devono tenere all'interno di quest'Aula. Con questo, le facciamo tanti auguri per questo suo nuovo incarico. Siamo sicuri, vista la sua professionalità, che lo

Presidente, la ringrazio per aver voluto svolgere questo suo intervento, che poi, ovviamente, non poteva non suscitare, da parte dei Gruppi, analoghi sentimenti e valutazioni, molto rapidamente, come deve essere nel costume dell'Aula e come la dottoressa Serafin per prima suggerirebbe, secondo la sua attenta attività di custode e interprete delle regole del Parlamento. Questi attimi di apprezzamento e di stima sono rivolti al futuro che la la dottoressa Serafin avrà, in un incarico importante in una società importante, di quelle che rendono l'Italia protagonista sui mercati internazionali, ma anche per ringraziarla di tutta l'attività che ha svolto, non solo da Segretario Generale. In precedenti legislature, anche non da senatore, ma da membro del Governo, ho potuto apprezzare la pazienza e la costanza con cui, non ancora Segretario Generale, dirigeva e coordinava i servizi dell'Aula. Ci sono persone alle quali estendo l'apprezzamento e la stima rivolti alla dottoressa Serafin; al dottor Toniato, che ha assunto l'incarico in una successione naturale dovuta all'esperienza e al lavoro svolto, e a tutti i Vice Segretari che sono stati designati. Vedo il dottor Sassoli che consente un regolare funzionamento dei lavori dell'Assemblea con una grande maestria. Si tratta di persone che fanno funzionare il Senato, il Parlamento, la democrazia e la Repubblica che, nonostante gli insulti alle istituzioni, costituiscono il fondamento e il baluardo della democrazia e della libertà. Grazie alla dottoressa Serafin e a chi oggi continua questa opera perché aiuta a far funzionare

dottoressa Elisabetta Serafin, che voglio ringraziare davvero di cuore a nome di tutto il Gruppo Partito Democratico. La dottoressa Serafin è stata una Segretaria Generale che ha accompagnato

alcuni dei quali ci sentiamo ancora - la dottoressa Serafin ha dimostrato di essere terza, imparziale e di mettere al centro della sua azione l'interesse di Palazzo Madama. È quello che auguriamo sempre ai prestatori d'opera e ai *civil servant*, come lo sono tutti i lavoratori del Senato e di tutti gli altri organi costituzionali. Mi permetterà, Presidente, di farle un in bocca al lupo di cuore, perché quarant'anni di vita qui dentro non sono una parte della vita, ma la vita nella sua interezza, certamente quella professionale. Non sappiamo e lei non saprà mai come sarebbe stata la sua se avesse scelto Banca d'Italia. Dalla sua biografia ha avuto un bivio nella vita tra la Banca d'Italia e il Senato. Ha scelto il Senato; sicuramente la sua vita è stata un po' più movimentata, di là sarebbe stata forse un po' più regolare e meno dentro alcune dinamiche che poi hanno fatto la storia della Repubblica. In bocca al lupo di cuore, dottoressa Serafin. Magari avremmo avuto la prima Governatrice della Banca d'Italia, chi lo sa?

avevamo previsto e non perché i Presidenti dei Gruppi di opposizione si cimentino in operazioni di chiromanzia, siamo arrivati al bivio finale, ministra Casellati. Oggi è previsto da calendario il completamento della discussione generale

la maggioranza non c'è. La maggioranza ha deciso di non presentare emendamenti. Avevo creduto alle parole del presidente Gasparri quando ci siamo scontrati più volte in questi passaggi non semplici, che ci hanno portato al completamento della discussione generale, ma è accaduto in Aula esattamente quello che era accaduto in Commissione: la maggioranza, signor Presidente, non c'è.

lavorare insieme per evitare danni alla nostra Costituzione, per evitare che fratture insanabili poi non possano essere ricomposte, non aver trovato nemmeno un emendamento di tutti i Gruppi di maggioranza ci fa prevedere prevedere una non semplice navigazione nella fase successiva alla discussione generale. Per queste ragioni, signor Presidente, per evitare che i

perché la maggioranza ha deciso anche di disertare il confronto politico in Aula, non presentando nessun emendamento. In questa condotta noi leggiamo una volontà netta, chiara

in discussione generale - di fermarvi, perché la disponibilità delle opposizioni al confronto nel merito c'è tutta. Alla vigilia dell'ultimo scorcio di discussione generale,

alcune decine di migliaia di persone. Le chiedo, per favore, di ascoltare quello che sto per dire e vorrei chiedere un'informativa urgente. C'è una situazione - lei lo starà leggendo - che è quella che è: la terra che trema in maniera molto significativa, purtroppo, da molte settimane a questa parte. Siccome capita che oltre a tremare la terra tremano pure le popolazioni, mi sembrerebbe il caso che l'Assemblea del Senato - naturalmente anche quella della Camera, ma quello lo decideranno loro - si potesse, nel corso delle prossime ore, occupare di questo, perché c'è una situazione obiettivamente di grande tensione e di grande preoccupazione su un territorio peraltro molto popolato le chiedevo la parola esclusivamente per questo. dobbiamo cercare di rispondere evitando tutte le conseguenze che si possono evitare, cioè quelle evitabili.

per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica***

che - lo dico subito - è ampia tanto quanto hanno chiesto tutte le forze politiche che - lo ricordo - hanno comunque presentato oltre 3.000 emendamenti. È iscritta a parlare la senatrice Rossomando.

Prima che prenda la parola, vorrei rinnovare il cordoglio di tutto il Senato per il lutto del suo caro papà, che ci ha fatto sentire ancora più vicini alla nostra Vice Presidente.

moltissimi interventi dell'opposizione e in particolar modo del mio Gruppo; aggiungerò alcune parole, alcune considerazioni, anche se il campo è stato già molto arato. Si è denunciato lo scambio che è avvenuto nella maggioranza sulle tre riforme di autonomia differenziata, premierato e giustizia; vorrei dire che non c'è solo l'obiezione su quanto sia censurabile nel metodo questo tipo di approccio, che tradisce perlomeno la noncuranza con cui si approccia un argomento delicato come quello delle riforme sull'assetto istituzionale.

scardinamento di tutta l'architettura della nostra Costituzione. Qui interviene un primo punto della discussione, anche pubblica, che ancora è in atto: non si tratta di contrapporre conservatorismo costituzionale a un approccio di innovazione, di riforme. È stato detto che non è che non si può toccare la Costituzione. Io vorrei dire una cosa con grande convinzione, cioè sgombrare il campo da un equivoco di fondo; poi confrontiamoci, ovviamente, però diciamo con estrema chiarezza che non si vogliono fare delle riforme della Costituzione, ma si vuole riscrivere la Costituzione, si vuole riscrivere la storia che ha condotto alla scrittura di questa Carta costituzionale e lo si capisce molto chiaramente nella lettura di queste tre riforme insieme. L'architettura della nostra Costituzione si basa su alcuni principi, alcuni dei quali alcuni dei quali sono l'equilibrio e la dialettica, il pluralismo che è stato menzionato, cioè la dialettica tra i poteri dello Stato. E questo è un punto che viene messo in discussione e travolto dalle riforme che vi apprestate ad approvare. Si basa anche su una democrazia partecipativa, sul pluralismo e sulla rappresentanza. Tutto questo, cioè la dialettica tra i poteri dello Stato, viene sostituita dal cosiddetto *Premier* pigliatutto, nel senso che il Presidente del Consiglio è un capo regolatore di ogni cosa; un capo affidatario. Alla dialettica parlamentare e alla dialettica tra i poteri dello Stato che sono alla base delle democrazie liberali viene sostituito un capo affidatario, con un'unica occasione di incontro con la volontà popolare, che è il voto (l'unico voto che potranno esprimere i cittadini, votando direttamente il Presidente del Consiglio). Certo allora che si poteva riformare e non mancavano ovviamente modelli a cui ispirarsi, perché di soluzioni ne abbiamo offerte noi delle opposizioni (valga per tutte il modello tedesco, con il rafforzamento delle competenze del Parlamento in seduta comune). Quei modelli quelle proposte non mettevano in discussione la dialettica tra i poteri dello Stato, né l'equilibrio e il ruolo del Parlamento. L'altra questione su cui bisogna sgombrare il campo è che c'è una domanda a cui vengono date risposte sbagliate, non so se intenzionalmente o meno. La domanda di stabilità non sta nell'accentramento dei poteri in una sola persona, nella mortificazione del Parlamento e nella disarticolazione dell'equilibrio tra i poteri, perché un altro principio che viene attaccato è quello della rappresentanza: non aver sancito chiaramente quale sarà la soglia minima per il premio di maggioranza, infatti, com'è stato ribadito più volte, comporterà una serie di conseguenze che scaturiscono da un unico fatto concreto,

un cenno all'autonomia differenziata: oltre a tutti i problemi già evidenziati per le enormi sperequazioni che cresceranno nel Paese, avremo

a prescindere dalle questioni giudiziarie, credo che le cronache di questi ultimi mesi dovrebbero farci molto riflettere su questo. Vi sono quindi un'integrale riscrittura dei poteri dello Stato e dei loro rapporti e una concezione verticistica del potere unita al mito del capo pigliatutto, che sarà in grado di controllare - grazie all'investitura popolare e al controllo sulla sua maggioranza - ripeto, sulla sua maggioranza gli altri poteri dello Stato, per arrivare fino al Presidente della Repubblica, che - vorrei ricordarlo ancora una volta - ha un ruolo sempre *super partes*, di mediatore tra i poteri dello Stato e di garante ultimo della Costituzione e dell'unità nazionale. Anche qui, Anche qui, le cronache politiche internazionali ci suggeriscono che proprio questo tipo di figura del Presidente della Repubblica, così come in Italia, è quello che più garantisce anche una convivenza pacifica e una ricomposizione dei conflitti in senso alto e in senso politico, perché, laddove chi ha tutti questi poteri è rappresentante di una sola parte, vediamo che i conflitti non si compongono, con una serie di crisi gravi del sistema. Nella vostra riforma, il Presidente della Repubblica, sia nella fase della sua elezione, quanto nello svolgimento del mandato, inevitabilmente sarebbe fortemente condizionato dal Presidente del Consiglio e dalla sua maggioranza. E ancora, poi ai contrappesi. Entro un certo arco di tempo, ovviamente, a questo punto avremo un Presidente della Repubblica politicamente omogeneo alla maggioranza di Governo e la nomina di ben dieci giudici costituzionali, che sono una questione importantissima nel controllo tra i poteri e nell'equilibrio, potrebbe avvenire nell'orbita politica e culturale della sola maggioranza parlamentare. [**Presidenza del vice

quindi chiaramente, di nuovo, la maggioranza politica sarebbe sovra-rappresentata in un organismo che rappresenta un punto di equilibrio. Per non parlare del progetto di far diventare il CSM un organo assolutamente burocratico. Insomma, stiamo parlando di queste tre riforme, che sono in realtà - come dicevo - una riscrittura della Costituzione. È di fatto un progetto accentratore e autoritario. Qui non interessa assolutamente discutere di richiami al passato o alle ideologie del passato. I fatti parlano, sono chiari e inequivocabili. Abbiamo fatto delle proposte e non una di tali proposte ha trovato non dico l'accoglimento, ma neanche la vostra attenzione. Proprio sul piano dei pesi e contrappesi, abbiamo proposto di di innalzare i *quorum* per eleggere i Presidenti delle Camere e gli organismi di garanzia e abbiamo avanzato proposte sul rafforzamento del Parlamento in seduta comune.

non so se questo risultato, che è assolutamente inequivoco e inequivocabile, sia stato voluto sin dall'inizio e corrisponda a una visione, che in realtà è teorizzata anche in altre parti d'Europa, di superamento delle democrazie liberali. Sta di fatto che il risultato sarà questo. a quanti in questa maggioranza si appellano spesso all'idea di libertà e ai principi liberali: ma davvero vi riconoscete in questa riforma? Ma davvero vi sentite legati, quando si tratta di cose così importanti, al vincolo di maggioranza? Davvero non ritenete di dare un contributo costruttivo? Davvero non ritenete di dover alzare la voce in un momento così importante? Noi possiamo

quando la presidente del Consiglio Meloni si è presentata in quest'Aula per chiedere la fiducia del Senato, io mi astenni e precisai che avrei avuto un animo aperto, con riserva di valutare provvedimento per provvedimento. A questo criterio mi sono attenuto e a questo criterio mi atterrò anche oggi. Anzi, in questa materia credo che l'animo particolarmente aperto sia particolarmente necessario. Io condivido due obiettivi fondamentali di questa riforma: una maggiore governabilità e una maggiore stabilità dei Governi, due obiettivi ovviamente collegati. Ma sono contrario alla proposta che ci viene presentata, perché credo che sia controproducente rispetto agli obiettivi stessi che si propone e che condivido. A mio parere questa riforma ridurrebbe la governabilità dell'Italia, anziché accrescerla, e fallirebbe proprio nel suo obiettivo centrale. Renderebbe praticamente e direi volutamente impossibili i Governi di larga collaborazione, di unità nazionale. Ci sarà pure una ragione se il Parlamento, non sondaggi di opinione o la stampa dei poteri forti, che forse una volta c'erano, hanno approvato con le più elevate percentuali di fiducia la nascita di tre Governi di unità nazionale: uno presieduto dal sottoscritto, con l'88 per cento dei voti del Parlamento, per fronteggiare la crisi finanziaria;

tre gravi crisi molto diverse (la tipologia delle crisi può includerne anche altre), un eminente politico e due non politici chiamati a guidare il Paese con larghissime coalizioni. Che cosa avrebbe fatto in quei momenti un *Premier* eletto da una maggioranza di parte e quindi legittimato a governare con la parte sconfitta alle elezioni, tendenzialmente vocata a fare opposizione? Con un Presidente della Repubblica che non potrebbe neppure esortare a fare uno sforzo di unità e con un *Premier* che magari, essendo venuto meno il *Premier* vittorioso alle elezioni, è entrato in carica sotto il vincolo di rispettare il programma di governo presentato alle elezioni dal *Premier* venuto meno, programma forse di due o tre anni prima, di valore ormai archeologico? Si può proporre una tale Costituzione in una fase storica che potrebbe vedere l'Europa e l'Italia in guerra tra qualche mese? L'Europa e l'Italia di nuovo in una grave crisi finanziaria, speriamo un po' più in là, e forse l'Italia in condizioni di lotta sociale nelle strade e nelle piazze, se continuerà la caduta senza speranza del salario reale? Ecco, proporrei di guardare avanti e vorrei anche rivolgermi a coloro che hanno certamente più sensibilità politica di me (magari potranno riconoscermi una certa esperienza nell'aver provato situazioni nelle quali nessuno dei presenti e pochissimi italiani dall'inizio della storia della Repubblica si sono trovati). Mi rivolgo ai politici, per i quali ho un grande rispetto, e a quanti ritengono che il premierato riavvicinerebbe i cittadini alla politica. Io temo che questo sia un drammatico errore di prospettiva. Oggi - lo dico con dolore la politica, i politici, non solo in Italia, riscuotono poco rispetto, tanto sospetto e molta diffidenza. In questa riforma i nostri concittadini vedranno il tentativo corporativo di chiudere ogni piccolo varco che permetterebbe, ove necessario, alla società civile di dare un suo contributo alla soluzione dei problemi del Paese. Devo dire con una punta autobiografica che, quando mi sono presentato davanti alle Camere per chiedere la fiducia, in una situazione esposta ad alto rischio di fallimento per il Paese, avevo due soli elementi di conforto oltre alla fiducia del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: l'aver avuto l'aver avuto l'88 per cento del Parlamento a sostegno di questa ipotesi di Governo e ancora di più il fatto che tutti sapessero che non mi ero certo candidato io per fare questo compito. Sarebbe stato enormemente presuntuoso. Non so con quale coraggio un candidato *Premier* diventerà tale sapendo che possono capitare queste sfide, e i cittadini naturalmente avranno il diritto di pensare che quella persona si ritiene la migliore in Italia in grado di far fronte ai problemi del Paese. Stiamo attenti che quello che magari viene pensato per avvicinare, non venga invece visto negativamente dai cittadini, i quali possono dire: tengono chiuse le corporazioni, grandi o piccole, dai tassisti ai concessionari balneari, e adesso vogliono chiudere anche la politica

concittadino europeo Macron, amato o detestato da molti, ma che certamente ha un'autorevolezza molto maggiore di quella che potevamo avere nel 2011 noi poveri chiamati dell'ultimo momento per risolvere una situazione, ha impiegato sei anni per fare una riforma delle pensioni, pur con l'autorevolezza del Presidente della Repubblica francese, ed ha avuto spargimento di sangue nelle strade. Ebbene, non sono più i tempi che hanno entusiasmato molti di noi, quelli che ricordo anch'io quando ero studente, ossia quelli della Repubblica presidenziale americana e della Repubblica presidenziale francese. Oggi abbiamo un sistema molto più duttile e vogliamo mandarlo al macero? Concludo, signora Presidente. La maggioranza vittoriosa del 2022 ha valorizzato il concetto di Nazione. Proprio perché ho grande rispetto per questo concetto e soprattutto per la realtà della nostra Nazione, l'Italia,

di una graduale frammentazione di fatto della Nazione in ogni dimensione possibile: la geografia istituzionale, con l'autonomia differenziata; la frammentazione sociale, con un sistema fiscale che prende ai meno abbienti per dare ai più abbienti, fondato com'è su regressività e condoni; come risultato di questa eventuale riforma, la frammentazione politica, che cristallizzerebbe la divisione e non la cooperazione, il reciproco disprezzo e non la disponibilità a collaborare, sino al voler rendere impossibile il lavorare insieme anche in momenti di possibile grave emergenza per la nostra Nazione.

ci tenevo ad essere qui oggi, perché a me pare che chi svolge una funzione parlamentare e ha l'onore di svolgerla in questa legislatura può mancare a qualche dibattito ma non a quello probabilmente più importante e più delicato,

Certo, mi si dirà che è la politica: dobbiamo bruciare i tempi; abbiamo bisogno di usare questo argomento forte in una imminente e importante campagna elettorale. Quale dimostrazione più chiara e lampante della strumentalizzazione? Se si fa di una discussione così delicata, così importante - almeno su questo siamo d'accordo, è delicata - perché incide profondamente negli assetti costituzionali, se la si usa come un qualunque argomento di battaglia politica, allora siamo nel pieno della strumentalizzazione. Probabilmente il ragionamento è stato questo: il Governo, il primo Governo a guida di una *leader* politica di destra, non accompagnato e sdoganato, come è stato il presidente Fini dall'esperienza di Berlusconi, ma in prima persona, facendo molta difficoltà sul terreno economico e sociale, prova a portare a casa, per il proprio popolo, per la propria gente, altri "ossi". la Lega, quella che è stata definita purtroppo, felicemente o infelicemente, secessione dei ricchi. Poi, una riforma della giustizia che è finalmente, per alcuni, una mordacchia ai giudici. Infine, per quello che Piero Ignazi ha definito, efficacemente, il "polo escluso", la possibilità di mettere una firma alla Costituzione, di riscriverne una parte. Una Costituzione che è stata vissuta, per alcuni, anche come uno schiaffo in faccia, perché partorita dalle grandi forze democratiche

Questa maggioranza, in questa esperienza di Governo, avrebbe dovuto fare l'esatto contrario: sfidare chi oggi è all'opposizione e si è anche misurato col Governo proprio sul terreno delle politiche sociali, sulla vita materiale delle persone; fare una legge sul salario minimo e magari poi rinfacciarci che la si è fatta durante questa legislatura e non in precedenza; fare una grande operazione sulla sanità pubblica, che possa rispondere ai bisogni dei cittadini e farli sentire meno soli, ad esempio quando debbono rinunciare alle cure. fare un avanzamento sulla base dei diritti, soprattutto dei diritti delle donne e delle giovani generazioni. Poi, sì, contemporaneamente, sfidare le forze politiche tutte a preparare una legislatura costituente; quello sì avrebbe messo in difficoltà, nell'uno e nell'altro caso, chi oggi svolge una funzione di opposizione. Questo avrebbe richiesto, ovviamente, innanzitutto uno spirito costituente o almeno uno spirito riformista. A me piace ricordare i lavori dell'Assemblea costituente, perché lì il dibattito sulla figura del Presidente del Consiglio, quindi sull'articolo 95, fu articolato e dialettico. Se ne occupò innanzitutto la sottocommissione sui problemi costituzionali, concentrando in particolare il dibattito sull'analisi comparata con gli altri sistemi costituzionali europei e internazionali. Questa Commissione fu il luogo di dibattito tra giganti del costituzionalismo, come Tosato e Mortati, da una parte, Terracini e La Rocca, dall'altra: i primi convinti che fosse necessario riservare al Capo del Governo un ruolo costituzionale autonomo, capace di imprimere all'esecutivo una direzione univoca,

e, io direi, per fortuna, fu preferita quest'ultima opzione, affidando al Presidente del Consiglio un ruolo di *primus inter pares*: una scelta netta e anche piuttosto peculiare nel panorama del diritto pubblico comparato; figlia, certamente, anche della traumatica esperienza fascista e di un certo senso di sfiducia riservato al potere esecutivo, che solo pochi anni prima era stato lo strumento per la distruzione della nazione e la disgregazione della comunità nazionale. Ma non fu solo questo il motivo, la ragione di fondo di un'opzione costituzionale di questa portata: valorizzare la collegialità del Governo, custodire il valore del massimo equilibrio tra i poteri dello Stato, affidare in ultima istanza al Presidente della Repubblica il ruolo di garanzia: ciò rende la nostra Costituzione il capolavoro politico istituzionale riconosciuto e ammirato nel mondo. Un'ispirazione ideale, politica e giuridica che deve continuare a guidarci, ancora oggi e ancor più di fronte al progetto di riforma che siamo chiamati a discutere, che sarà un nuovo *unicum*. Io non so se gli attuali neo costituenti siano più alti d'ingegno dei Padri costituenti, se siano più capaci, se abbiano intuito meglio. Poi, qualora malauguratamente, dovesse questa riforma diventare un fatto, magari diventerà l'esempio nel mondo.

stravolgendo assetti e confini dell'architettura istituzionale. L'onorevole Terracini metteva in guardia i colleghi dal pericolo che l'eccessivo rafforzamento della figura del Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe finito per autorizzare quest'ultimo: «a *fare la politica di un partito della coalizione**,* anziché quella *della coalizione* nel suo complesso», nonché «dalla circostanza di dare eccessivi poteri ad uomini che avrebbero potuto non meritarlo». Sul secondo pericolo preferisco non esprimermi, sebbene abbia una chiara opinione sul fatto che questo Governo e chi lo guida non meritino affatto un potere tanto indefinito. Sul primo punto, invece, ritengo sia opportuno fermarsi perché rappresenta il cuore stesso delle criticità del progetto che ci viene presentato. D'altronde il premierato nasce esattamente per questa ragione: un riassetto del potere esecutivo completamente affidato alla figura del *Premier*, che è anche *leader* del partito di maggioranza relativa e dunque detentore assoluto della guida del Governo e della supremazia del Parlamento. Davanti a tutto questo è incredibile notare come, quasi ottant'anni prima, i Padri costituenti avessero previsto, come testimoniano le dichiarazioni appena citate, il rischio di degenerazione che è all'ordine del giorno del nostro dibattito pubblico e dei lavori parlamentari odierni. Una degenerazione evidente e innegabile che passa per lo svuotamento del ruolo del Parlamento e per la mortificazione delle funzioni di garanzia in capo al Presidente della Repubblica, custode dell'unità nazionale e della tenuta democratica del Paese. Se questa riforma vedrà la luce, ci ritroveremo catapultati in un sistema costituzionale senza termine di paragone possibile tra quelli internazionali. Un caso unico di concentrazione del potere nelle sole mani del *Premier* che, unito al progetto di autonomia differenziata in discussione, determinerà uno stravolgimento del sistema Paese per come lo abbiamo conosciuto in settanta anni di storia, come spiegato prima ma benissimo dalla senatrice Rossomando. La nostra contrarietà netta e senza appello rispetto rispetto a tutto questo è già stata ampiamente espressa nei mesi che abbiamo alle spalle. Lo abbiamo fatto e continueremo a farlo e lo faremo non perché siamo pregiudizialmente contrari ad un confronto sulle riforme persino di rango costituzionale, pur non ritenendole - voglio sottolineare - la necessità prioritaria del Paese, il quale invece ha bisogno di inverare ancora molte indicazioni della Carta costituzionale che sono rimaste

anche sul merito dell'idea di riorganizzazione dei poteri dello Stato, dal sistema tedesco a una nuova legge sui partiti, su cui non torno. Quella che il Governo e la maggioranza ci propone, ignorando ogni proposta e ogni tentativo di confronto, è invece un'avventura, una sperimentazione unica al mondo, un ircocervo istituzionale. Quest'Aula ha ascoltato le parole sagge e autorevolissime della senatrice Liliana Segre che voglio ricordare: «Anche le tribù della preistoria avevano un capo, ma solo le democrazie costituzionali hanno separazione dei poteri, controlli e bilanciamenti, cioè gli argini per evitare di ricadere in quelle autocrazie contro le quali tutte le Costituzioni sono nate». Possiamo dire con forza che l'Italia non ha bisogno di una "capocrazia", come nel titolo del felice libro di Michele Ainis, ma soprattutto non vuole sprofondare nella preistoria della cultura giuridica, politica e costituzionale alla quale questa riforma pericolosa ci condurrebbe.

E allora il mio consiglio, Presidente, emerge da alcune carte che sono conservate in Senato, patrimonio dell'archivio del Senato della Repubblica. Mi riferisco al materiale relativo alla Fondazione del Movimento Sociale Italiano che contiene molte cose interessanti a partire da una lettera ad Alcide De Gasperi. C'è scritto come nasce quel partito, perché si chiama Movimento Sociale Italiano e qual è il rapporto con la Repubblica sociale italiana,

perché altrimenti, invece che togliere ogni sospetto, lascerete ogni speranza, sarete sempre quelli che vengono da lì e tornerete presto ai margini.

con il suo permesso e con un po' di pazienza da parte dei colleghi, vorrei raccontare una storia agghiacciante, ma a lieto fine. fine. C'era una volta e c'è ancora in Europa un Paese che quando era una nostra provincia si chiamava Britannia, capitale Londinium. Un Paese che ha un regime istituzionale decisamente incredibile, se non fosse vero. In quel Paese si vota mediamente una volta ogni cinque anni e si elegge un capo, un vero capo, perché quell'eletto, che in quel Paese si chiama *Prime Minister*, si trascina con sé il Governo,

Può sciogliere il Parlamento senza chiedere il permesso al Presidente della Repubblica, che lì si chiama *King* o *Queen*, può cambiare i Ministri quando egli decida che non servono più al loro scopo e se per caso nascesse qualche conflitto istituzionale, come spesso accade nei Paesi democratici, in quel Paese non c'è nemmeno una vera e propria Corte costituzionale, anzi, per non farsi mancare niente, non c'è nemmeno una Costituzione scritta. Aggiungo che quel capo eletto ha i cordoni del bilancio che si fa consegnare dal Ministro delle finanze in una celebre, consunta valigetta in marocchino rosso la quale lui, Presidente del Consiglio, o meglio *Prime Minister*, presenta al Parlamento, il quale non ha nemmeno la possibilità di emendare. La regola è guardare ma non toccare. C'è di peggio: a questo capo, tramite un organismo *ad hoc*, fanno riferimento i pubblici ministeri, i quali, neanche a dirlo, sono separati dai giudici e non hanno la obbligatorietà dell'azione penale. Mamma mia,

il Re non ha neppure il potere della *moral suasion.* Il Primo Ministro gli scrive un discorso, il Re si presenta in Parlamento, lo legge, e ha soltanto la capacità e la volontà - è questo l'unico potere che gli rimane - di dire: «*My Government*», come se fosse il suo Governo o ne avesse fatto parte o avesse scelto lui qualche cosa, invece niente, è uno spettatore. Ho detto che si trattava di una storia terribile, la storia di un tiranno, la storia di una tribù preistorica, ha un lieto fine, perché quei britannici, grazie a una rivoluzione nel 1688, si inventarono questo sistema. Si inventarono i partiti politici, costrinsero il Re nei limiti dei poteri del Parlamento e si vaccinarono per secoli. Si vaccinarono contro l'assolutismo, contro il giacobinismo, giacobinismo, contro Napoleone che esportava il giacobinismo con le baionette; si vaccinarono contro il comunismo, contro il fascismo, contro il nazismo e vinsero dandoci, assieme ai loro giovani allievi americani, la nostra libertà. *(Applausi)*. Ecco la storia di un capo tribù preistorico. La ricordo per dire, cari colleghi, che il premierato non è il regime della tribù, è una forma di democrazia come altre e la Britannia è lì che lo testimonia.

Il Partito Democratico dimentica anche la storia della Francia, della riforma De Gaulle, la quale fu all'inizio censurata più volte per anni come autoritaria, se non fascista, salvo poi scoprire che era cosa buona e giusta e fonte di salvezza il giorno in cui un socialista nel 1981 si inventò un campo largo e vinse le elezioni. Il Partito Democratico si dimentica anche della storia e della Costituzione tedesca, che pure richiama il modello del premierato, perché quando si arriva al nodo del modello del cancellierato, che oggi il Partito Democratico propone, il nodo, il perno, cioè il potere di scioglimento in capo al cancelliere, il Partito Democratico lo salta a piè pari: il modello tedesco è un modello mezzo tedesco. Sarà perché il tedesco è una lingua difficile, ma fino là non ci sono arrivati. Agli amici dei 5 Stelle, con i quali ho con simpatia interloquito tante volte durante i mesi del lavoro nella Commissione affari costituzionali, vorrei dire vengo loro incontro. Il Parlamento è schiacciato dal Governo con tutti quei marchingegni che conosciamo, non da questa legislatura: li conosciamo da venti o trent'anni, lasciatevelo dire da uno che ha purtroppo tanti anni. È schiacciato, sempre con molta simpatia vi vorrei chiedere, cari amici, se andava meglio quando si potevano sospendere le libertà costituzionali con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri all'ora dei telegiornali della sera? Oggi noi siamo orgogliosi di celebrare i settantasei anni della nostra Costituzione, ma ecco un caso unico al mondo:

Conoscete la storia, ogni tanto l'avete citata: i tentativi di modificare la Costituzione furono iniziati ben prima che la Costituzione entrasse in vigore, nel 1948, perché i Padri costituenti temevano proprio la deriva assemblearista, il controllo dei partiti, i poteri forti e così via. Tentativi di riforma erano stati fatti in numero enorme; Antonio Malaschini lo scorso anno ha pubblicato uno studio in cui mette tutti in fila questi tentativi di riforma e li commenta. A questo proposito, siccome ho nominato un ex Segretario Generale, ne approfitto per fare i miei auguri e congratulazioni al nuovo Segretario Generale. *(Applausi)*. Dal 1981 (tentativo Spadolini) al 2016 (tentativo Renzi) passano trentacinque anni: vi ricordo i tentativi di modifica della Costituzione su questo punto dei poteri del Presidente del Consiglio e del Governo, passano attraverso i nomi di Speroni, De Mita, Maccanico, D'Alema, Berlusconi, Napolitano e Letta (ce n'è qualcuno di sinistra in questo elenco, vero?).

mai successo che, in questo tentativo di rafforzamento dell'Esecutivo, qualcuno obiettasse che andavamo verso l'uomo brutto, nero e cattivo, la tribù. Obiezione: questo testo del Governo però è difettoso. Lasciatemelo dire con onestà, al meglio di me: se l'obiezione è tecnica e non è pretestuosa o pregiudiziale, sono disposto a discuterne e ad accoglierla, perché effettivamente problemi in questo testo ancora attualmente ce ne sono. Del resto, chi per primo disse e sollevò queste obiezioni sul testo fu il Presidente del Senato, in primo luogo, e il presidente della Commissione affari costituzionali, senatore Balboni, in secondo luogo, poi altri. Di cambiamenti e modifiche ne sono stati fatti in Commissione, a dimostrazione che forse la maggioranza stava silenziosa, ma lavorava. Ora, ci risiamo: se dovessi riconoscere le incongruenze del testo, direi che ce ne sono. sono. Ad esempio, è pleonastico il voto di fiducia dopo le elezioni del Primo Ministro: se il popolo l'ha eletto oggi, domani non è necessario che raccolga la fiducia dal Parlamento. Dico anche che altre incongruenze ci sono e riguardano, ad esempio, la mancanza o l'aggiunta di contrappesi, che potrebbero essere maggiori. Vi è la mancanza dello Statuto dell'opposizione, che peraltro non lo vuole, perché aveva votato contro, e così via, ce ne sono altre. Se però dovessi racchiudere le mie riserve e le mie obiezioni su questo testo, direi che c'è un punto che è importante: il testo di riforma dice che

Molte cose sono rimandate a una legge elettorale: con molta onestà, franchezza, critica e autocritica, vi dico che non tutto si può fare mediante una legge elettorale, senza una previsione costituzionale che le dia un sostegno.

Si può fare con la sola legge elettorale? Cosa accade se i poli elettorali politici invece di due sono tre? tre? Cosa si fa con il premio di maggioranza: a quale soglia lo fermiamo? Ecco che sono dubitoso che tutto questo si possa fare con la sola legge elettorale e avrei preferito che si fosse lavorato di più sul testo della Costituzione.

prendano nota e possano modificarlo. Però questo vuol dire che dobbiamo lavorare ancora un po'. Vuol dire cioè, che il testo non è chiuso. Ci sarà la possibilità di emendarlo in quest'Aula? Me lo augurerei. Temo di no, purtroppo, lo confesso. Me lo augurerei. Ci sarà la possibilità di modificare nell'*iter* successivo il disegno di legge? Bisognerà che ci sia, perché altrimenti il testo rischia seri problemi di costituzionalità.

dei problemi che ci sono: meglio affrontarli. Dobbiamo soltanto avere paura della nostra paura, e cioè di evocare il rischio e le tenebre del capo della tribù preistorica.

Presidente, colleghe e colleghi, carissimo Ministro,

Cerco di rilevare due modalità di espressione, senza mettere l'uno contro l'altro. Io odio il calcio balilla della politica: ci si fa male e basta;

e l'intervento astioso, un pochettino pessimistico, del senatore Monti, campione mondiale di non essere mai stato eletto, ma di aver avuto garanzie per tutta la vita per quello che avrebbe fatto. Beato lui, dico io, o forse sfortunatamente questo Vede, Presidente, questo provvedimento legislativo nasce in un momento particolare di disaffezione della gente a partecipare al voto; un periodo tragico, anche per come è stato gestito, della pandemia. Ma soprattutto avviene in quest'Aula, dove noto, essendo anziano - anzi, meglio, vecchio l'opposizione nelle parole, ma anche nella comunicazione non verbale, ha vinto il campionato mondiale di acredine, di sospettosità, di doppiopesismo, di evocazione di tragedie orribili, partendo da un punto per me estremamente negativo: la sfiducia totale nel popolo. Ma come? Il popolo italiano, con tutti i difettucci, è meraviglioso. Ha saputo ricomporsi dopo la guerra. Ha saputo ricomporre, almeno in parte, riscrivendo in parte la storia, le ferite, anche tra fratelli, di tanti anni. Ha saputo reagire a Tangentopoli. Ha saputo reagire alla messa al confine di un *Premier* forte ed importante. Ha saputo reagire al terrorismo; in epoche recenti, alla pandemia e a tanti malgoverni. Ha reagito con dignità, qualche volta con contraddizione, ma sempre in maniera encomiabile. È un popolo buono, è un popolo che vuole la pace, non solo contro le guerre degli altri, ma anche nelle guerre locali, quelle della delinquenza organizzata, alle quali stiamo reagendo.

all'innovazione, partendo da un punto fondamentale: la fiducia nel voto del popolo? Come si fa a dire che il popolo ci porterà allo scatafascio? Ma che pensate della gente, quella gente che lavora, quella gente che spera nel lavoro, quella gente che ha reagito alla pandemia, quella gente che ha reagito - cari colleghi - a troppi troppi ordini dall'alto di Presidenti del Consiglio non votati, con provvedimenti liberticidi? Stiamo scherzando o stiamo cercando di evocare una realtà difficilmente accettabile e contenibile? Noi vogliamo dare fiducia alla gente, che deve essere responsabile di quello che vota. Dobbiamo dare fiducia al futuro *Premier*, che, assumendo con enorme responsabilità il potere di decidere in parte in una democrazia reale, non può non sentirsi coinvolto in maniera fondamentale nella sua coscienza e nei suoi atti. Abbiamo un popolo che deve essere più responsabilizzato - e così sarà - e un confortato dalle elezioni del popolo, potrà lavorare meglio. Basta: non si evoca nessuna tragedia, nessuna azione muscolare dal Presidente della Repubblica e dal Capo del Governo. Ma stiamo scherzando? Di che cosa stiamo parlando?

gente ha prodotto l'integrazione scolastica delle persone con disabilità, la chiusura degli ospedali psichiatrici e ha reagito senza panico, ma con molta sofferenza, alla pandemia che ci ha portato a essere un po' tutti, in maniera assolutamente ingiustificabile, prigionieri di noi stessi. Eppure siamo andati avanti a testa alta - ripeto - con qualche contraddizione, perché siamo italiani. Siamo contemporaneamente uniti da alcuni ideali, da alcune idee e dalla storia e divisi da un po' un po' di diversità, che però ci fa bene, se la accettiamo come valore e non come peso. Della diversità italiana e tra gli italiani io sono orgoglioso *(Applausi)*, essendo - se mi permettete,

con cose sacre laicamente. Apriamo le porte al nuovo, perché così chiede la storia, così chiede la società civile oggi. La paura o, peggio, il ricatto di vedere il male solo negli altri e il bene solo in noi noi ci ha fatto male troppe volte. Questo doppiopesismo, sì, è pericoloso per la democrazia: la delegittimazione delle idee degli altri. Signora Presidente, con molta umiltà, sono molto felice di partecipare positivamente al voto per il premierato, anche perché ne condivido i modi, partecipati per lungo periodo, e ne concepisco positivamente i contenuti.

nella fiducia delle persone e di chi sanno consapevolmente, dignitosamente, liberamente eleggere,

scommettere sul futuro sapendo che sta nelle buone mani delle persone.

da nessuno che sono astiosamente contrario al premierato. Io sono del tutto favorevole a modifiche sostanziali nel nostro sistema elettorale e, quindi, anche alla elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma non posso non sposare la tesi espressa qui dal presidente Monti, ossia che non è con questa legge che noi facciamo il miglior servizio alla nostra democrazia. Al presidente Pera, con tutta la simpatia che nutro per lui, ricordo però che in Inghilterra gli eletti in Parlamento sono rappresentanti dei rispettivi collegi elettorali, non della Nazione in senso lato come prevede la nostra Costituzione. E ricordo che in Inghilterra, quando un Ministro viene accusato di aver commesso il seppur minimo reato, si dimette immediatamente, cosa che qui da noi non succede. *(Applausi)*. Signora Presidente, uno dei mantra ripetuti fino allo sfinimento dai componenti dell'attuale maggioranza è il seguente: noi le promesse elettorali le manteniamo. La promessa fatta era di eleggere direttamente il Presidente della Repubblica oppure il Presidente del Consiglio per rendere più stabile il quadro politico e governare meglio il Paese. Quindi l'obiettivo dichiarato è la stabilizzazione del quadro politico. Prima di decidere come mantenere questa promessa, sarebbe opportuno riflettere sul perché si è arrivati alla situazione attuale. Ricordiamo tutti quello che è successo nel nostro Paese dopo il superamento del Mattarellum, che era un sistema elettorale attorno al quale era nata la Seconda Repubblica, e non aveva solo il merito di promuovere il rapporto tra eletto e territorio attraverso i collegi uninominali, ma aveva anche alla base un forte fondamento maggioritario che spingeva i partiti a organizzarsi su una logica bipolare. Il Porcellum e l'Italicum, oltre al mostro delle liste chiuse, hanno invece favorito la frammentazione dell'offerta politica, senza prevedere alcun meccanismo correttivo in grado di garantire a chi vinceva le elezioni una maggioranza per poter governare. E da qui nascono tutti i problemi dell'oggi: il fatto che i cittadini non scelgono gli eletti, le maggioranze mutevoli, i Governi ballerini e i *Premier* non in linea con la volontà popolare. Finché i meccanismi elettorali hanno favorito stabilità e alternanza, il sistema, con tutti i suoi limiti, ha funzionato. Quando, però, le regole sono diventate pasticciate, il sistema si è inceppato. E poteva incepparsi anche due anni fa, quando siamo stati eletti noi. Andate a rileggere le proiezioni sui seggi del Senato. Se le opposizioni non si fossero spezzate in tre tronconi, bastava un accordo tra centrosinistra e terzo polo, per non dire tra centrosinistra e MoVimento 5 Stelle, e in quest'Aula la destra non avrebbe avuto la maggioranza. maggioranza. Io speravo che la Presidente del Consiglio, consapevole di tutto questo, di avere goduto di un contesto particolarmente favorevole, ne tenesse conto nell'attuare l'impegno programmatico, assunto dalla sua parte politica, di rendere più governabile il Paese. che di questo si sta parlando: di rendere più governabile il Paese. Come farlo, modificando la Costituzione, rivedendo le leggi in essere o tutte e due, ne è la conseguenza. Certo, la suggestione di cambiare la Costituzione è stimolante e probabilmente è foriera di un maggior consenso di parte. Ma è davvero la cosa migliore per l'Italia e per chi ci vive? La Costituzione fu scritta con il contributo di tutte le forze politiche elette, il 2 giugno 1946, nell'Assemblea costituente. Non avrebbe avuto più senso, nel solco di quell'esperienza, un patto con le minoranze per scrivere una legge elettorale in grado di coniugare governabilità e rappresentanza? E poi un intervento minimo, tra Costituzione e Regolamenti parlamentari, per imprimere al sistema elementi di stabilità, con l'introduzione, per esempio, della sfiducia costruttiva? Invece, si è scelta una strada completamente diversa, con un intervento tanto invasivo quanto semplicistico - mi si consenta di dirlo - sul cuore della Costituzione. Non basta dire che questo faceva parte del programma elettorale. Lo ha spiegato bene il senatore Franceschini: la maggioranza ha tutto il diritto di avanzare questa proposta, ma, quando si interviene sulla Costituzione, non si può non mediare con le opposizioni. Conosco l'obiezione: in Commissione avete pazientemente ascoltato le nostre proposte. Peccato, però, che non ne abbiate accolta una. Allora, questo non è ascoltare: è sentire, che vuol dire fingere di ascoltare. Trovo poi, piuttosto volgare e di comodo insinuare che, con questa riforma, la sinistra, per andare al Governo, dovrà vincere le elezioni. I Governi che si sono succeduti in questi anni sono legati al fatto che nessuna coalizione aveva i numeri in Parlamento e, da qui, tutti sono andati al Governo: la Lega, che nel 2018 di certo non aveva vinto le elezioni, rompendo, tra l'altro, il vincolo di coalizione; la stessa Forza Italia, che ha sostenuto sia il Governo tecnico di Mario Monti, che quello di Mario Draghi, che la nascita del Governo di larghe intese con Enrico Letta.

Come a dire: ora che siamo in maggioranza, la cambiamo noi la vostra Costituzione nata sulle ceneri della Resistenza, notoriamente poco gradita da questa parte politica, dalla vostra; la Costituzione, quindi, come uno scalpo, per riscattare una storia di presunta esclusione di alcuni dirigenti e di una parte di certo non maggioritaria dell'attuale elettorato di centrodestra. Lo scalpo sta proprio nel colpire i pesi e i contrappesi del nostro sistema elettorale e le ragioni storiche che ne sono alla base, che sono però le ragioni che l'hanno reso impermeabile, finora, a qualsiasi torsione autoritaria. Da qui una riforma che rende il Presidente del Consiglio, da *primus inter pares* di un organo esecutivo, *dominus* assoluto del sistema, sulla scorta di una legittimazione che passa non più dal Parlamento, ma da un atto plebiscitario. Va bene, ma forte di un sistema che, nei fatti, introduce il vincolo di mandato per i parlamentari. Il Presidente del Consiglio avrà un potere di interdizione assoluto circa l'elezione dei Presidenti di Camera e Senato, del Presidente della Repubblica, dei giudici costituzionali e dei membri laici del CSM. Il *quorum* deliberativo dei tre quinti potrebbe essere raggiunto anche senza confronti complessivi con l'opposizione, grazie all'aggiunta, con legge, di pochi parlamentari della maggioranza e del Governo. tutte questioni sollevate da diversi costituzionalisti in questi mesi, che però non hanno convinto la maggioranza proponente a integrare la norma con elementi di bilanciamento. E per non farsi mancare nulla non si è voluto rinunciare all'impronta populista, cancellando i senatori a vita, senza pensare al ruolo che questi senatori di nomina presidenziale hanno avuto nella storia del Parlamento, del contributo che hanno portato e che continuano a portare su questioni di scienza, di memoria storica e sul valore delle istituzioni. Quel che è peggio, Presidente, è che questa riforma toglie alla nostra democrazia uno degli elementi di maggior pregio, ossia la capacità delle istituzioni di reggere e assorbire qualsiasi crisi. Certo, questa capacità è stato spesso mal usata e ha dato vita a fenomeni di trasformismo che occorreva sradicare; ma, per farlo, si è cucita una camicia di forza che ossifica le istituzioni introducendo regole inutilizzabili davanti a crisi o minacce. Ognuno ha la sua idea sugli accadimenti della storia repubblicana, ma cosa sarebbe successo con queste nuove regole tutte le volte che il Paese è andato in crisi e ha avuto bisogno di stringersi attorno ai valori dell'unità e della solidarietà nazionale? Con questo premierato l'interruttore di sicurezza sarebbe stato e sarà in futuro una nuova campagna elettorale che, anziché unire, dividerà ancora di più il Paese. La verità, Presidente, è che con questa riforma il popolo non decide nulla, ma ha la possibilità di indicare ogni cinque anni chi dovrà decidere al suo posto. Il potere è concentrato in una sola persona scelta dalla maggioranza di coloro che votano. I precedenti del passato inquietano. Questo provvedimento è l'apoteosi del modo di questa destra di fare politica con la p minuscola, quella che fa l'interesse proprio e dei "propri amici" e non della comunità nazionale nel suo insieme. È inevitabile che, per vincere le elezioni, si faccia propaganda; ma, quando poi si governa, continuare a fare propaganda crea danni enormi non solo al Paese, ma soprattutto alla nostra democrazia, perché passa l'idea che essere "amici" di chi governa conviene. Credete davvero che gli italiani non si renderanno conto che questa non è una riforma, ma è l'ennesima bandiera propagandistica da agitare in vista delle elezioni europee? È un obiettivo miope, signori, e di breve periodo, anziché lungimirante quale dovrebbe essere una Costituzione. Noi a questo disegno non ci stiamo perché il prezzo da pagare, non per il Governo o le opposizioni, ma per la nostra democrazia rischia di essere altissimo. Siamo in una fase storica nella quale le democrazie sono sotto attacco. lo sono anche in Europa dove assistiamo alla nascita delle "democrature", cioè a sistemi democratici nella forma, ma autoritari negli aspetti sostanziali. Che l'Italia possa mettersi sulla scia di tutto questo è un rischio che non possiamo assolutamente permetterci. *(Applausi)*. PRESIDENTE.

noi siamo preoccupati del tono e del taglio con cui questo dibattito si sta sviluppando. E assistiamo con una certa qual preoccupazione al fatto che da destra e da sinistra si stia approcciando a un percorso così elevato, significativo e pesante per una democrazia quale la riforma della Costituzione, con toni che vanno a metà strada fra la ricerca spasmodica di legittimazione, da un lato, e la crociata, dall'altro. Come non definire altrimenti un dibattito nel quale la nostra Presidente del Consiglio ha definito questo lavoro che ci accingiamo a compiere, anzi, che stiamo già compiendo, la madre di tutte le battaglie, rievocando - non so quanto consapevolmente - una frase il cui *copyright* è di un dittatore iracheno che la coniò nel momento in cui doveva lanciare una guerra. E credo che le metafore belliche dovrebbero, soprattutto di questi tempi, essere utilizzate con grande parsimonia, attenzione e cautela. e cautela. Questa presunta riforma che sarebbe la madre di tutte le battaglie o di tutte le riforme, che dir si voglia, non fa altro che tradire un'ansia di legittimazione da parte di una *Premier* che in sé probabilmente ha la consapevolezza di essere stata, sì, legittimata dal voto degli italiani e dal consenso del Parlamento, ma al tempo stesso di essere stata legittimata da una maggioranza relativa degli italiani o, se preferite, da una minoranza superiore ad altre minoranze. E ciò avviene tenuto conto del fatto che le elezioni del settembre del 2022 hanno visto la singolare circostanza per la quale le attuali opposizioni al Governo Meloni si sono presentate divise fra loro, ma la somma dei loro rispettivi consensi è stata superiore rispetto a quelli raccolti dalla coalizione guidata dalla *premier* Giorgia Meloni, la quale, evidentemente sente dentro di sé un'ansia da legittimazione che la spinge già oggi a commettere un primo errore politico significativo. quello di chiudere la discussione, il dibattito, il confronto e rimandare già al *referendum*, come una sorta di lavacro finale di legittimazione totale, l'intero percorso. In questo In questo senso, le parole del senatore Pera sono state una sorta di messa in mora di questa riforma; un avviso ai naviganti per chi ha la consapevolezza di udire cosa ha significato tra le righe, ma neanche troppo, una personalità così autorevole: l'obiettivo

e cioè il fatto che, a fronte di un errore di impostazione muscolare da parte della destra, corrisponde un errore di impostazione da parte dell'opposizione - o meglio di buona parte di essa - che sceglie da subito i toni della crociata, immaginando di sfidare la maggioranza non tanto sul piano dei contenuti riformisti, quanto invece sul piano della contrapposizione dialettica in maniera alternativa, a prescindere dai contenuti di merito. Ebbene, crediamo che il Paese, e quindi conseguentemente il Parlamento, si debba sottrarre a questo spettacolo e questo lo pensiamo, signora Presidente, perché abbiamo l'ambizione di poter rappresentare all'interno di queste Aule quella vocazione riformista che è sempre esistita nel nostro Paese, che nei passaggi fondamentali ha saputo dare voce anche ad alcuni momenti significativi e rischia di essere compressa, negletta o silenziata di fronte al doppio spettacolo muscolare cui facevo riferimento in precedenza. Tra che all'interno del mondo composito - repubblicano, progressista - del centrosinistra esistano diverse vocazioni non è scoperta di oggi e non è neppure scoperta solo del nostro Paese. è stato citato prima, che credo sia interessante, perché la storia è sempre maestra di vita e chi non la studia non sa da dove arriviamo e di conseguenza, con grande difficoltà può immaginare di portarci verso l'avvenire. Mi riferisco al dibattito che avvenne in Francia all'indomani della grande crisi che quel Paese visse a seguito della crisi di Algeria, una crisi che consentì a quel Paese di dotarsi di istituzioni che regolano il meccanismo repubblicano. Noi, signora Presidente, abbiamo vissuto un parallelo come quello della crisi di Algeria a cavallo dell'inizio degli anni Novanta. E siamo ancora qui a discutere adesso su come dobbiamo ammodernare le istituzioni, su come dobbiamo riformare il sistema, su come bisogna essere all'altezza di corrispondere ad una lettura in cui il popolo si senta rappresentato dalle istituzioni. Ebbene, in Francia, nel 1956 e negli anni seguenti, ci fu un bel dibattito che contrappose - da un lato - François Mitterrand, che guidava quella che noi oggi potremmo definire la sinistra radicale, e - dall'altro lato - Maurice Duverger, che guidava un percorso di sinistra riformista e che arriverà addirittura ad essere europarlamentare nel 1989 eletto nelle liste del Partito Comunista Italiano (per dire la composizione di una realtà molto composita dal punto di vista della dialettica). Duverger nel 1956, contrapponendosi a Mitterrand, che supportava la tesi della proporzionale pura che aveva determinato la crisi della Quarta Repubblica, sosteneva l'introduzione dell'elezione del Primo Ministro e arrivò a dare il proprio consenso al sistema semipresidenziale come surrogato rispetto all'idea del premierato. Qual era la tesi? Tra la confusione e l'ordine democratico, è sempre meglio l'ordine democratico. Io credo che questi elementi dovrebbero dirci qualcosa. Come dovrebbe dirci qualcosa una rapida carrellata delle esperienze che ci sono state sul tema specifico dell'elezione diretta del Primo Ministro in quel in quel mondo riformista a cui facevo riferimento in precedenza. All'inizio degli anni Novanta, in corrispondenza di quella crisi, davanti all'assurdità delle forze politiche dell'epoca, le Associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI) lanciarono una campagna nella società civile per rilegittimare e superare la crisi, per una migliore qualità della democrazia. Per iniziativa di un senatore dell'epoca, il senatore De Matteo, venne presentato un disegno di legge per l'elezione diretta del Primo Ministro. Ma noi vorremmo anche legarci in maniera ancora più intima e strutturale nel nostro percorso alla tesi n. 1 dell'Ulivo, che è stata forse la pagina forse la pagina più significativa, la più alta, più preziosa del riformismo italiano, che al proprio *incipit* parlava del Governo del Primo Ministro e proponeva l'indicazione del candidato *Premier* da parte del corpo elettorale, introducendo nel proprio programma una convenzione costituzionale per giungere allo scioglimento del Parlamento e all'indizione di nuove elezioni in caso di cambiamenti di maggioranza. Peraltro, questi temi vennero ripresi, uno per tutti, da Mario Segni e da un composito e articolato gruppo di parlamentari repubblicani, liberali, democristiani dell'epoca, presentando il 22 luglio 1993 un disegno di legge costituzionale per l'elezione diretta del Primo Ministro e del Presidente della Regione. Peraltro, questo tema fu esattamente al centro dei lavori della Commissione bicamerale per le riforme

nel quale, quando qualcosa viene presentato dal presidente D'Alema, diventa improvvisamente sacro ed intangibile, come il Talmud o come le tavole del Sinai; quando viene proposto da qualcuno che non va a genio al presidente D'Alema e ai suoi epigoni, diventa improvvisamente un'eresia della quale non si può neppure più parlare. Eppure noi vorremmo proseguire in questo solco, magari riprendendo anche quanto inserito nella proposta di legge costituzionale dell'allora deputato Franco Monaco - prima che venisse affetto da una particolare sindrome di antirenzismo - che aveva proposto, nel gennaio del 2003, scartando il semipresidenzialismo e il cancellierato, la necessità di introdurre il modello del premierato e la scelta premierato e la scelta fondamentale, cioè quella di consentire agli elettori l'elezione contestuale del Presidente del Consiglio dei ministri e della sua maggioranza. Mi verrebbe da dire che noi staremmo sulla logica del Franco Monaco del 2003 e meno sulle sue più successive conversioni sulla via di Damasco. Il punto è quindi che, ribadita l'esigenza di affrontare in maniera laica, riformatrice, di merito la nostra discussione, tutto questo dibattito rischia di essere inficiato da un punto qualificante, che è anche il contenuto degli ordini del giorno il contenuto degli ordini del giorno G1 e G2, che mi appresto ad illustrare, che dal nostro punto di vista diventano la cartina al tornasole rispetto alla qualità di questo lavoro e anche alla volontà reale della maggioranza, la quale è stata sfidata in diversi interventi rispetto alla buonafede dietro la quale si teme che non esista invece una reale volontà riformatrice.

all'esame e all'approvazione della nuova legge elettorale. Ora la maggioranza, se ha davvero a cuore la bontà del processo riformatore, ha l'occasione per dimostrare su questi ordini del giorno che è possibile trovare una strada che non sia la contrapposizione muscolare o, peggio ancora, l'utilizzo della riforma della Costituzione per la finalità di una raccolta di facile consenso. Perché diciamo questo? Dobbiamo Dobbiamo ricostruire la dimensione identitaria della nostra Repubblica, che Scoppola aveva definito la Repubblica dei partiti e che vedeva e ha visto per tutta la cosiddetta Prima Repubblica un piano trascendente, che subordinava e in qualche misura scavalcava anche le Aule parlamentari rispetto al luogo della decisione (oggi si direbbe della sovranità e dell'esercizio della democrazia). Qual era questo luogo trascendente? Erano le sedi dei partiti di Governo e del principale partito dell'opposizione. Oggi discutiamo a lungo del ruolo e della natura del Presidente della Repubblica: ci siamo già scordati che nel 1978 il presidente della Repubblica Leone diede le dimissioni semplicemente perché una delegazione di partiti si presentò al Quirinale e gli disse la direzione della DC, il comitato centrale del Partito Comunista e la direzione del Partito Socialista avevano deciso che se ne doveva andare a casa? E quel Presidente della Repubblica se ne andò a casa senza neppure convocare una discussione parlamentare nella quale si entrasse nel merito della questione. Ecco, quella era la natura della Prima Repubblica, nel bene e nel male, che è stata travolta, cambiata, modificata e strutturalmente rivista all'indomani della crisi del 1992-1994, ma che non ci ha posto nella discussione per poter costruire un meccanismo equilibrato all'indomani di quella crisi. crisi. La legge elettorale che fu introdotta allora - con il sistema maggioritario - imponeva inevitabilmente una rivisitazione del sistema del bicameralismo perfetto, che non accadde; imponeva naturalmente l'introduzione dello Statuto delle opposizioni, che non venne fatto; imponeva un'armonizzazione del nostro sistema rispetto a quella modifica, connaturata con l'elemento strutturale. Ora ci troviamo di fronte a una novità ulteriore: questa riforma propone sostanzialmente di introdurre nella Carta costituzionale l'elemento maggioritario. In origine era addirittura sancito con il 55 per cento dei seggi assegnati; ora, dopo una discussione in sede di Commissione, si è stabilito di togliere una cifra, ma si è stabilito di sancire il meccanismo del premio. È inevitabile quindi che ci siano due elementi che devono precedere questa discussione: il primo è che tipo di legge elettorale ci vogliamo dare e il secondo è la rottura del meccanismo del bicameralismo perfetto. Diversamente lo voglio ribadire una volta di più alla signora Ministra e lo dico ai colleghi - ci state presentando una proposta che apparentemente andrebbe a rafforzare la governabilità, ma che in realtà costruisce una ragnatela per qualsiasi *Premier* che dovesse essere eletto. Egli verrebbe, infatti, imprigionato dal meccanismo del bicameralismo perfetto del bicameralismo perfetto e dalla logica del cosiddetto diritto di fronda, avendo mantenuto al proprio interno il meccanismo sulla base del quale un secondo *Premier* può sostituire in corso d'opera e con voto parlamentare quello eletto direttamente dai cittadini. Non ci vuole molto a capire

la polemica stucchevole tra un Vice *Premier* che ha proposto di reintrodurre la leva obbligatoria, un altro Vice *Premier* che invece ha detto che non se ne parla, perché non ci sono i soldi, e il Ministro della difesa, che ha detto che assolutamente non bisogna farlo. *(Applausi)*. Ecco, immaginiamoci se questo stile dovesse essere applicato alla nuova riforma costituzionale, con un Vice *Premier* che farebbe campagna elettorale per sé in Parlamento, assicurando che non scatterebbero le prerogative dello scioglimento, nel caso di una sostituzione in corso d'opera. Capite perché è indispensabile che ci sia un percorso di questa natura? E poi, naturalmente, la questione che rimanda alla legge elettorale rimanda all'esigenza, cari colleghi, di ridefinire il ruolo, la natura, la funzione del sistema dei partiti nel nostro Paese. Se non componiamo questo mosaico contestualmente con gli altri tasselli, oltre alla vicenda del premierato, premierato, rischiamo di fare un vestito strappato, una situazione monca. Se non affrontiamo finalmente e fino in fondo la natura dell'applicazione dell'articolo 49 della nostra Costituzione, per dire che cosa sono oggi i partiti, come si fa il processo nella formazione della politica e della partecipazione dei cittadini all'interno di questo tipo di strumenti, che tipo di democrazia interna essi hanno, che tipo di statuti devono avere per corrispondere effettivamente ai contenuti della nostra Costituzione, se non affrontiamo questo nodo, continuiamo a permanere nell'equivoco di fondo, anche con riferimento alle polemiche di questi giorni sul finanziamento pubblico e sulla possibile reintroduzione del finanziamento dei partiti. Se non definiamo la natura dei partiti e continuiamo a rispondere in termini emergenziali, continueremo a rimanere all'interno di questo limbo infinito della transizione italiana. La seconda questione è quella a cui facevo riferimento in precedenza: abbiamo già presentato un emendamento per chiedere la rottura del bicameralismo perfetto. Lo diciamo in particolare alla maggioranza. Se volete perseguire davvero e coerentemente la questione dell'autonomia differenziata (lasciamo stare il merito e stiamo alla questione funzionale), se davvero credete all'autonomia differenziata, serve in maniera essenziale una Camera che presidi il meccanismo legislativo dell'autonomia differenziata. *(Applausi)*. Non possiamo avere un sistema in cui le due Camere fanno lo stesso mestiere per i poteri residuali dello Stato e poi l'equilibrio fra i Governatori e il *Premier* eletto è affidato a una dinamica vertenziale tra il Primo Ministro e il Governatore di turno. Non è così che si realizza una democrazia compiuta; quindi è inevitabile che si affronti e che si vada lungo questo percorso sulle questioni di armonizzazione. Il nostro ordine del giorno - mi avvio alla conclusione, signora Presidente - va esattamente nella direzione che ho cercato di descrivere. C'è una bella C'è una bella frase di Mahler, che ci ispira e sulla quale vorremmo cercare di convincere gli altri colleghi. Una frase secondo la quale la tradizione non è il culto delle ceneri, ma è la custodia del fuoco. Se sostituiamo alla parola "tradizione" la parola "riformista", ci sentiremo tutti a casa; ma, se noi sostituissimo alla parola "tradizione" la parola "democrazia", noi vorremmo che ci sentissimo tutti davvero qui dentro a casa.

sono mesi che sentiamo parlare, in questo Parlamento e in quest'Aula, di autonomia differenziata e di istituzione del premierato, per affrontare e dare una soluzione all'instabilità politica. Ora, io vorrei che le parole che diciamo abbiano un senso e che tra di noi ci capiamo. Ci rinfacciate tutti i giorni che questo è un Governo politico e dite all'opposizione

per indebolire il Parlamento e il Capo dello Stato. Questo è chiaro. Dopodiché si possono fare tanti marchingegni e si può discutere di mille cose; però quello che voi proponete e che state facendo è esattamente questo.

se avessimo affrontato con la stessa determinazione e lo stesso tempo la questione della crisi energetica, della crisi climatica o del precariato,

non vedono un grande futuro rispetto alle cose che stiamo facendo e questo produrrà - sì - degli effetti devastanti, se non affrontiamo questi temi in termini molto determinati e urgenti. Questa discussione Questa discussione sul premierato non dà alcuna risposta a questi temi. Che, risposta dà alla questione ambientale o alla questione climatica, che vediamo tutti i giorni? Che risposta dà alla crisi economica alla crisi economica delle persone? Si dice che sono aumentati gli occupati: vero dal punto di vista numerico, però sono diminuite le ore lavorate, è diminuito il reddito dei lavoratori e delle lavoratrici, i giovani fanno fatica a trovare un posto di lavoro e ad avere una prospettiva per il futuro.

Questo è il dato. Anche con la proposta del Governo D'Alema, che fu approvata, non abbiamo risolto i problemi di questo Paese; anzi, anzi, è sotto gli occhi di tutti che cos'è diventata la sanità nel momento in cui è stata regionalizzata. Siamo di fronte al fatto che le persone fanno fatica a curarsi, fanno fatica a trovare una soluzione rispetto ai loro problemi. Quindi, avrei capito come fare una discussione insieme per capire dove si è sbagliato, che cosa introdurre e come correggere. Questo è il dato fondamentale. Però qui c'è un rovesciamento della Costituzione del 1948, nata dalla lotta partigiana e antifascista.

da tutti. Questo è il dato fondamentale: era una Carta costituzionale condivisa, perché la democrazia è una fatica, costruire democrazia vuol dire cercare di ascoltare, capire, includere e non

davvero: pensate che aumentiamo la partecipazione dei cittadini se neghiamo il ruolo, ad esempio, delle forze sociali, che sono gli elementi che stanno nella società e che dovrebbero partecipare? Pensiamo che ridurre i partiti a macchine elettorali risolverà questo problema? Penso di no, perché sempre meno gente va a votare. Perché questo accade? Perché quello che dicono, che pensano e che vivono viene poco ascoltato, anzi non viene rappresentato.

perché è il *Premier* che trascina ed è tutto nelle sue mani, a questo punto sarà molto difficile che io faccia una discussione critica nei suoi confronti: questo è il dato fondamentale. Per questa ragione

se loro non partecipano alla politica, comunque quest'ultima fa delle scelte che ricadono su di loro, quindi è necessario ricostruire una rappresentanza che sia la più proporzionale possibile, in modo che tutti si sentano rappresentati.

per rispondere con altrettanta simpatia al presidente Pera. Colgo l'occasione anche per ringraziarlo per il lavoro svolto in Commissione e per aver ravvivato con i suoi interventi in discussione, anche con le sue proposte formulate per iscritto, una Commissione affari costituzionali che da parte della maggioranza altrimenti sarebbe stata veramente da elettroencefalogramma piatto. D'altra parte, anche oggi i banchi vuoti della maggioranza, che purtroppo non sono inquadrati (perché viene inquadrata l'oratrice), dimostrano davvero l'assenza totale e il disinteresse della stessa maggioranza per una proposta di riforma costituzionale potenzialmente deflagrante. presidente Pera, però devo sottolineare che i parallelismi non sono il suo forte. Mi permetta di dirlo, perché ha paragonato la democrazia italiana e il sistema italiano, che è un sistema giovanissimo, con un sistema, quello della Gran Bretagna, che invece è probabilmente il più antico del mondo. Già nel 1215 si diede la *Magna Charta Libertatum*, che limitava i poteri del sovrano. Nel 1600 cominciano a nascere i primi partiti politici; nel 1649

della Gran Bretagna. Questo è un primo parallelismo. L'altro parallelismo che lei sbaglia è quando paragona i DPCM usati dal presidente Conte in piena pandemia, per arginare un'emergenza sanitaria di livello globale, che non si era mai affrontata prima, con i DPCM che invece voi utilizzate in legge di bilancio per definire i LEP, i livelli essenziali di prestazioni nell'autonomia differenziata, che non è un'emergenza. Quindi, vi arrogate un diritto e un potere, quello sì strabordante, strabordante, utilizzando in maniera distorta uno strumento che va usato *cum grano salis*, come lo usò il presidente Conte in piena pandemia. *(Applausi)*. Mi dispiace dover fare questo appunto, però ho trovato una caduta di stile in questo paragone. D'altra parte, lo stile non è esattamente ciò che caratterizza questa maggioranza. I greci la chiamavano *hybris*. In termini moderni, mutuati dalla psicanalisi, si chiama, invece, delirio di onnipotenza. È quella tentazione a cui nessun uomo, oggi, sa resistere; purtroppo, sembra che possiamo aggiungere: neanche alcune donne. È la sensazione, quando la fortuna e il successo arridono loro, di sentirsi così forti e così fortunati da cedere alla tentazione di dare l'assalto al cielo. Lo abbiamo visto, d'altra parte, già accadere in precedenza, con il conferenziere d'Arabia, con l'incantatore di cammelli, Matteo "*Mehmet"* Renzi, quando, reduce del suo 40 per cento alle europee del 2014, tenta anche lui l'assalto al cielo e propone la sua riforma costituzionale, l'*all in* e dicendo di giocarsi il tutto per tutto. Dopo gli italiani scopriranno che, naturalmente, bluffava e rimaneva abbarbicato alla mensa della politica, ma tentò anche lui l'assalto al cielo. Come sempre capita a chi è preda di *hybris*, cadde miseramente, per non rialzarsi mai più; e dall'idea di fare il "Sindaco d'Italia", passare a fare il sindaco di Riad è stato un attimo. però, dai precedenti storici, che avrebbero dovuto insegnarvi qualcosa, non avete invece imparato nulla e vi siete fatti guidare proprio dalla *hybris*, dal delirio di onnipotenza, seguendo cioè per questa riforma costituzionale gli appetiti e gli interessi dei singoli partiti; anzi, gli appetiti e gli interessi dei singoli *leader* *leader* di partito, anziché farvi guidare da quello che è il supremo interesse della nazione. Avete così dimostrato, appunto, di non aver imparato e avete generato un mostro informe: un sistema né presidenziale, né parlamentare, né zuppa, né pan bagnato, che non esiste in nessun altro luogo del mondo. L'aspetto divertente, in tutto questo, è che avete tentato anche di accollare la generazione di questo mostro a noi delle opposizioni. Andate ripetendo che, sì, è vero che nel programma elettorale noi avevamo promesso agli elettori il presidenzialismo; però poi, parlando con le opposizioni, abbiamo optato su questo premierato bifido, alla matriciana. Invece, no: no: la responsabilità è tutta vostra. Infatti, se voi pensate che promettere agli elettori il presidenzialismo e presentargli il premierato sia la stessa cosa, è perché non avete alcuna opinione del vostro elettorato e perché ritenete che non capiscano la differenza. Gli fate il gioco delle tre carte e pensate che non se ne accorgano. Allora noi decliniamo qualunque responsabilità in questo obbrobrio che voi avete sottoposto alle Camere che rappresenta l'ennesimo tradimento delle vostre promesse. Ricordo d'altra parte le le balle sulla rimozione delle accise, sul blocco navale, sulle pensioni minime a mille euro e sulla tassa sugli extraprofitti che vi siete rimangiati. Giorgia Meloni, quando era all'opposizione, diceva di voler abolire le Regioni; ora che è al Governo e potrebbe farlo, invece

poco cambia perché questo è come tenete in conto i vostri stessi elettori, che sono quelli che state ingannando. Questa modifica costituzionale è fondata su tre elementi principali: arroganza, falsità e negligente sciatteria. Naturalmente questi tre elementi sono tenuti insieme dal filo conduttore della volontà di riscrivere la storia dal secondo Dopoguerra ad oggi. Cominciamo dall'ultimo elemento, la sciatteria. La furia ideologica con cui avete impugnato una materia tanto delicata come quella della modifica costituzionale, che trasforma il nostro ordinamento istituzionale, si denota già nella forma in cui avete redatto il testo sottoposto alla Commissione. Non sia d'offesa a nessuno, ma il linguaggio utilizzato è più simile al linguaggio di un ufficiale del catasto, è certo lontanissimo dal linguaggio chiaro e perfetto che i nostri Padri e Madri costituenti utilizzarono nello scrivere la Costituzione. Già questo, di per sé, è uno sfregio alla Costituzione. lo dico io perché ricordo che il professor De Siervo, già Presidente emerito della Corte costituzionale, ha scritto nero su bianco, nelle memorie lasciate alla Commissione, che la qualità tecnica di alcune parti dell'originale proposta governativa appariva sconcertante. Qualità tecnica sconcertante. Poiché però la forma è strettamente collegata alla sostanza, vediamo come vi eravate presentati in Commissione. non c'era un tetto al numero dei mandati che il Presidente eletto poteva svolgere. In effetti è una dimenticanza da poco quando si va a normare l'elezione di una carica monocratica così importante. Vi era sfuggito? Non ci sconvolgiamo per questo perché c'è di peggio. Nella prima versione del testo che avete sottoposto alla Commissione avevate addirittura quantificato il premio di maggioranza, con un 55 per cento tondo tondo, scritto direttamente in Costituzione. Quando studiosi e osservatori trasversalmente, sia di destra che di sinistra, hanno mostrato perplessità, allora siete arrossiti e avete presentato i famosi quattro emendamenti del Governo. Governo. È comparso così un tetto al numero dei mandati; due, però due e mezzo perché è sempre meglio lasciarsi una scappatoia libera. Avete tolto inoltre il 55 per cento, ma lasciato il premio di maggioranza in Costituzione. in Costituzione. Il premio di maggioranza in Costituzione è l'aspetto più grave di questa riforma, è il pugnale conficcato nel cuore della Costituzione. Questo comunque avremo modo di dirlo più avanti. invece occupiamoci dell'altra sciatteria che avevate messo nel testo iniziale. Questa è bellissima; avete annunciato infatti *urbi et orbi* che uno degli obiettivi principali di questa riforma è quello di impedire i ribaltoni. E cosa avete fatto? Non solo con il vostro testo avete autorizzato il ribaltone, ma l'avete costituzionalizzato. Nel testo originale, infatti, voi avete scritto che in caso di cessazione della carica, il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare candidato in collegamento al Presidente eletto. Cioè sotto lo scranno del Presidente del Consiglio eletto avete piazzato una bella botola per farlo cadere e passare lo scettro direttamente al secondo in lista. fatto prima a scrivere che doveva incaricare direttamente Matteo Salvini, perché è chiaro che quella era una norma *ad personam*: forse una manina leghista nottetempo vi aveva inserito quel passaggio? Un pasticcio inverecondo, non si sa. Passiamo ora al testo attuale, quello che stiamo qui esaminando e che quindi ha passato il vaglio della Commissione dopo essere stato emendato dal Governo. Questa è la cosa più parossistica e tragicomica che c'è in questo testo. Dopo che vi abbiamo fatto notare questo piccolo dettaglio della botola, infatti, siete corsi ai ripari e abbiamo pensato che forse ci avevate pensato meglio e avevate fatto le cose per bene. Macché, peggio di prima, al punto che oggi è arrivato in Aula un testo in cui si dice che il Presidente della Repubblica può rinnovare l'incarico al Presidente del Consiglio morto. Ci siete arrivati fino all'Aula con un testo del genere, con una simile sciatteria, che davvero sembra un testo scritto dietro le quinte di «Zelig» anziché dentro le Aule di un Ministero. *(Applausi)*. State mettendo mano alla Costituzione, perbacco, un po' di serietà. Le falsità sono il secondo pilastro che sostiene questa riforma. Ce ne sono almeno quattro macroscopiche, poi ce ne sono altre minori che vedremo se avremo il tempo di illustrare.

con questa riforma sono i cittadini a scegliere chi li governa (con il sotto-corollario che ciò gioverà alla partecipazione alle urne), ed

Due balle al prezzo di una, perché non c'è alcun problema di governabilità e perché la Costituzione non c'entra un fico secco. Il Governo Meloni, infatti, detiene il *record* dei decreti-legge. In diciannove mesi ne avete emanati 61, a partire, come sempre ricordiamo, dal ridicolo decreto-legge in materia di *rave party* che, come si sa, è la peggiore piaga italiana, e avete posto 51 questioni di fiducia. Questo significa che il Governo Meloni viaggia ad una media di oltre tre decreti-legge al mese e quasi altrettante fiducie al mese. Chi è che sta impedendo al Governo Meloni di governare? Il Governo governa, eccome,

proprio la sua stessa maggioranza parlamentare, ridotta a fare la *claque*, ad essere una schiera di pigia bottoni plaudenti e inutili, come dimostrano anche in questa occasione in cui non hanno presentato neanche un emendamento sulla riforma costituzionale. Interpretate il vostro ruolo con un minimo di dignità. Se c'è un potere che ha bisogno di essere rafforzato, è quello del Parlamento, vera sede di rappresentanza del popolo e non il Governo o il Primo Ministro. Ve lo ha ricordato anche la senatrice Segre nel suo intervento della settimana scorsa, quando ha voluto stigmatizzare questa mistificazione e ha affermato: «Mi colpisce il fatto che oggi, di fronte alla palese mortificazione del potere legislativo, si proponga invece di riformare la Carta per rafforzare il già debordante potere potere esecutivo». È falso che il Governo non riesce a governare. E una balla è smontata. Passiamo alla seconda. Giorgia Meloni ripete ossessivamente di essere contraria ai ribaltoni e ai Governi tecnici e noi non potremmo essere più d'accordo. Del ribaltone che avete piazzato all'interno del testo della Costituzione già ho detto e quindi non mi ripeto. Ma c'è di più, perché anche qui mentite sapendo di mentire. Infatti, cari colleghi e care colleghe, i ribaltoni si contrastano - magari

modo si disincentiva questo malcostume tutto italiano contro cui noi del Movimento 5 Stelle ci siamo sempre battuti e siamo sempre stati solo vittime, mai artefici: noi non abbiamo mai accolto nelle nostre fila un transfuga, invece tutti tutti quanti voi non solo accogliete a braccia aperte voltagabbana, ma li andate anche a cercare, fate *scouting* - anche questo gli italiani lo sanno e se lo ricordano molto bene - addirittura promuovendo compravendite di senatori, come accadde sotto il Governo Berlusconi, con il noto scandalo del senatore De Gregorio e Valter Lavitola. Voi e i vostri alleati, che si sono dimostrati disposti anche a pagare milioni per cambiare i rapporti delle maggioranze, oggi volete passare da moralizzatori della politica? Avete preso gli italiani per stupidi, perché non c'è bisogno di cambiare la Costituzione per moralizzare la politica; sarebbe sufficiente averla una morale e agire di conseguenza. E un'altra balla è stata smontata. Vediamo un'ulteriore falsità, la più sottile, la più invisibile e quindi la più insidiosa. Voi dite, con un bello slogan confezionato apposta per ingannare la buona fede delle persone: decidi tu chi ti governa. Bello, è uno slogan efficace. Io vi chiedo chi è che fa le leggi, perché di fatto già adesso le fa il Governo, anche se dovrebbe farle il Parlamento. Abbiamo detto che avete varato 61 decreti-legge, il che non lascia materialmente tempo al Parlamento di legiferare, anche se gli fosse concesso, perché è sempre impegnato a convertire i decreti-legge. Chi li emana i decreti-legge? I Ministri. Allora, di fatto, oggi stanno già legiferando persone mai elette, perché Piantedosi, il Ministro dell'interno, non è stato eletto da nessuno, Abodi, Ministro per lo sport e i giovani, non lo ha eletto nessuno; Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito (qualunque cosa ciò significhi), Sangiuliano, il Ministro della cultura che premia libri che non legge, e Schillaci, Ministro della salute, chi li ha eletti? Nessuno, eppure sono loro che fanno le leggi per gli italiani. Questa è quindi un'altra balla che andate raccontando. Vediamo, dunque, in quale incubo vorreste trascinare l'Italia. Gli italiani e le italiane, secondo il vostro disegno, sono chiamati ogni cinque anni a votare e votano un Presidente del Consiglio che si trascina dietro un Parlamento servo, cui può staccare la spina in qualunque momento,

Mentite sapendo di mentire, perché voi state dando più potere a voi stessi, non agli elettori. E poco importa, come sarà davvero, come Giorgia Meloni va sbandierando in ogni dove, la legge elettorale, che ancora nessuno conosce e che tenete ben nascosta nel cilindro, per cui in questa sede stiamo ragionando di mezzo quadro, perché l'altra metà non ci è dato sapere come verrà composta. Poco importa se davvero metterete le preferenze nella legge elettorale, perché comunque saranno tutti burattini nelle mani del Presidente del Consiglio eletto, saranno tutti intercambiabili, tutti asserviti, perché nessun parlamentare vorrà che il Presidente del Consiglio stacchi stacchi la spina. Pertanto non cambia assolutamente nulla e non ci sarà nessuno che potrà impedire al Presidente del Consiglio di sciogliere le Camere per ragioni assolutamente imperscrutabili. Non ci sarà nessun controllo. Arriviamo al nodo della questione, all'inconfessabile cuore nero di questa riforma, il completo capovolgimento dei poteri. Quando l'Assemblea discuterà la nuova Costituzione, i banchi del Governo dovranno essere vuoti e, del pari, il Governo deve rimanere estraneo alla formulazione del progetto, se si vuole che quest'ultimo scaturisca dalla libera determinazione dell'Assemblea sovrana. Pietro Calamandrei, uno dei Padri costituenti, cioè uno che la Costituzione l'ha scritta. Certo, a leggere queste parole oggi viene quasi da sorridere di tenerezza, perché, pensate, chi ha scritto la Costituzione immaginava non solo che ogni modifica dovesse nascere nascere dall'Assemblea sovrana - noi, voi, noi - ma addirittura che il Governo non ci dovesse essere. E invece voi che cosa avete fatto per questa riforma costituzionale? La ministra Casellati, chiusa nel suo Ministero, ha confezionato un bel testo, che oggi il Parlamento è chiamato a ratificare. Ve lo ripeto: il fatto che non abbiate presentato emendamenti certifica la servitù a cui avete condannato il Parlamento rispetto al Governo, perché già vi comportate così e il premierato ancora non è stato approvato. Tale e tanto è lo spregio che avete per il Parlamento e per l'intero ordinamento dei poteri disposto dalla Costituzione repubblicana, che volete istituire un Parlamento completamente asservito al Capo del Governo, che detiene il potere di vita e di morte sulle Camere. Il Capo del Governo può cioè sciogliere le Camere come e quando meglio crede e questo lo fate vendendo agli italiani, nella vostra propaganda mistificatoria, il concetto di governabilità. Qui è la menzogna più grave: spacciate per una maggiore libertà dell'elettorato una modifica che assoggetterà il potere agli umori di una sola persona. È qui la pericolosità di questo disegno ed è qui la svolta autoritaria che caparbiamente vi ostinate invece a negare. È il contrario del diritto a partecipare, del diritto a contare e del diritto a essere rappresentati che voi sbandierate. Questa menzogna ne regge poi un'altra, molto interessante, ossia che l'elezione diretta del Premier farà anche da viatico contro l'astensionismo. Anche qui abbiamo due balle al prezzo di una, perché è facile constatare come nelle istituzioni e negli enti locali, dove già esiste l'elezione diretta del sindaco o del Presidente di Regione, ciò non abbia la minima influenza sulla partecipazione al voto. Questa infatti volete volete sapere come si fa ad incentivare? Vogliamo provare? La partecipazione al voto si favorisce con i comportamenti specchiati, che siano da esempio, contrastando la corruzione corruzione e candidando persone che non solo siano oneste, ma appaiano oneste. E invece voi chi candidate? Vittorio Sgarbi, indagato per riciclaggio d'opere d'arte. Difendete Santanchè, Ministra inquisita per truffa allo Stato. Vi arroccate tutti intorno a Toti, che pretende di governare una Regione dagli arresti domiciliari. Così pensate di incentivare la partecipazione al voto? E poi smantellate i presidi anticorruzione, cancellate gli strumenti d'indagine e mettete il bavaglio alla stampa e alla magistratura, verso la quale conducete una campagna diffamatoria e che volete addirittura sottoporre a perizia psichiatrica. La partecipazione alle urne si favorisce infondendo fiducia nelle persone verso la politica. Voi fate l'esatto contrario, perché vi va bene che vadano in pochi a votare: solo così vincete le elezioni. Infine, arriviamo al tormentone: non tocchiamo i poteri del Presidente della Repubblica. Repubblica. Da tutto quello che ho detto finora è evidente che il Presidente della Repubblica perde il potere di scioglimento delle Camere, così come quello di incaricare il nuovo Presidente del Consiglio eletto o di incaricarne un altro in caso di crisi. Voi sterilizzate la funzione del Presidente della Repubblica, lo pensionate da arbitro, lo declassate a spettatore e avete anche il coraggio di continuare a ripetere che però non toccate i suoi poteri. Ci vuole davvero una bella faccia tosta per ripetere questa falsità. State stravolgendo la Costituzione dalle fondamenta e vi ostinate invece a parlare di intervento chirurgico non invasivo. Ora, se davvero volessimo paragonarla ad un'operazione chirurgica, uso le parole di Nicola Grasso, professore di diritto costituzionale, dovremmo pensare a un intervento che sostituisce contemporaneamente i maggiori organi vitali, come il cuore, il cervello e i polmoni, con qualcosa di sicuramente incompatibile con l'assetto preesistente, che porterà alla sicura morte del paziente, ossia la nostra Costituzione repubblicana e i suoi principi e valori, che sono tenuti in piedi proprio dall'equilibrio dei poteri, che viene stravolto in questa riforma. Arriviamo alla fine di questo mio intervento. Avevo detto che questa riforma è fondata su tre pilastri: sciatteria (l'abbiamo vista), falsità e ora è il momento dell'arroganza. dell'arroganza. Vi leggo un brevissimo brano. La prima applicazione del premio di maggioranza in Italia (nella forma del *jackpot system*) si ebbe nel 1923, con l'approvazione della legge Acerbo (quella che aprì le porte alla dittatura fascista), che prevedeva l'assegnazione dei due terzi dei seggi della Camera dei deputati alla lista che avesse superato il 25 per cento dei voti. Nel secondo Dopoguerra, dopo un ritorno al sistema proporzionale, si reintrodusse il premio di maggioranza nel 1953, con la cosiddetta "legge truffa", in cui si prevedeva l'attribuzione di un premio in quota variabile alla coalizione che avesse preso la maggioranza assoluta dei voti validi. Non venne mai applicata, perché nessuna coalizione superò la metà dei voti, e fu abrogata. Nel 2005 è il turno della legge Calderoli, il noto Porcellum, di reintrodurre il premio di maggioranza in quota variabile. La legge Calderoli prevedeva l'assegnazione del premio alla singola lista o alla coalizione più votata, indipendentemente dal risultato elettorale. La Corte costituzionale l'ha ritenuta incostituzionale. La legge successiva è del 2015 e prevedeva anch'essa l'attribuzione di un premio di maggioranza a chi avesse superato il 40 per cento dei voti. Anche quest'ultima è stata dichiarata incostituzionale. Non vi ho letto un trattato di costituzionalismo, vi ho letto una pagina di Wikipedia. Neanche quella avete aperto per scrivere la riforma della Costituzione! *(Applausi)*. Nemmeno su Wikipedia avete guardato, perché altrimenti avreste saputo che tutti i precedenti storici nel nostro Paese di introdurre un premio di maggioranza o hanno aperto le porte alla dittatura oppure sono stati bocciati dalla Corte costituzionale, perché incostituzionali. Voi avete fatto peggio di Acerbo e del Porcellum messi insieme, perché almeno quelle erano leggi elettorali, che comunque sono leggi ordinarie. Voi lo mettete addirittura in Costituzione, ipotecando il futuro di questo Paese con un atto di imperio e di tracotanza senza pari, che gli italiani non vi consentiranno. Vado alla conclusione, perché, nonostante il tempo a mia disposizione fosse tanto, ci sarebbe da parlare del combinato disposto di questa follia con l'anarchia differenziata, un *mix* esplosivo esplosivo che, mentre sovverte i poteri, spacca il Paese. Veramente uno scenario da incubo, che non soltanto noi, ma gli italiani vi impediranno di attuare. Visto che è stata citata nuovamente in Aula poc'anzi, voglio rendere omaggio anche io alla senatrice a vita Liliana Segre, che, nonostante l'età, la settimana scorsa ha voluto essere presente e portare il suo contributo in quest'Aula. Con lo stile pacato che la contraddistingue, non ha però taciuto il suo grido di allarme e ha definito questa riforma una scelta avventurosa, aggiungendo non tutto può essere sacrificato in nome dello slogan "scegliete voi il Capo del Governo". Anche le tribù della preistoria avevano un capo, ma solo le democrazie costituzionali hanno separazione dei poteri, controlli e bilanciamenti, cioè gli argini per evitare di cadere in quelle autocrazie contro le quali le costituzioni sono nate. Ebbene, quello che Liliana Segre non ha potuto dirvi, perché compresa nella sua eleganza, ve lo dico io. Voi imitate le tribù della preistoria, perché è nelle grotte che siete rimasti ed è lì che volete trascinare nuovamente l'Italia. *(Applausi)*. Volete rendere l'Italia un Paese di cavernicoli, mai gli italiani avveduti ve lo impediranno.

Signor Presidente, inizio il mio intervento affermando sin da subito che condivido pienamente l'obiettivo di questa riforma. per noi, l'obiettivo principale di questa riforma è la stabilità del Governo.

si è trovato a svolgere il ruolo di parlamentare nelle ultime legislature, la XVII e la XVIII, in cui si sono susseguiti tutta una serie di Governi e di maggioranze che non sono emersi grazie a un voto chiaro, convinto e maggioritario degli elettori, ma per la necessità di formare dei Governi parlamentari. Ricordo che nella XVII legislatura il Partito Democratico e Forza Italia sono stati costretti a governare insieme, sostenendo Enrico Letta, che la legislatura poi è andata avanti, perché a fronte della sfiducia di Forza Italia e della sua uscita dal Governo, una sua parte, il Nuovo Centrodestra, ha deciso, senza rispettare il mandato elettorale, di sostenere un Presidente del Consiglio del Partito Democratico, Matteo Renzi; poi c'è stato il Governo Gentiloni.

formati da forze politiche che alle elezioni erano contrapposte e che sono state costrette, a causa di questo sistema imperfetto, a mettersi insieme pur di dare un Governo al Paese. Lo sappiamo tutti: il primo Governo Conte, sostenuto da Lega e 5 Stelle, il secondo da PD e 5 Stelle e poi il terzo, il Governo Draghi, in cui si sono unite gran parte delle forze politiche di quella legislatura. Quindi, è evidente a tutti che esiste un un problema di stabilità ed omogeneità delle forze politiche che hanno governato negli ultimi anni, a cui deve essere trovato un rimedio, una soluzione. Noi siamo convinti che fosse nostro dovere intervenire in questa legislatura per proporre una soluzione. C'è chi nel corso del dibattito ha fatto gli elogi del sistema tedesco, o del sistema anglosassone; io credo che non dobbiamo innamorarci di un sistema sistema o di un altro, ma dobbiamo individuare le singole soluzioni che possono migliorare il modello italiano, la Costituzione italiana Per raggiungere questo obiettivo, a nostro avviso, il sistema migliore che questa riforma introduce in modo chiaro e inequivocabile è l'utilizzo del premio di maggioranza. Il premio di maggioranza è l'unico strumento che permetterà di avere Governi di legislatura, Governi stabili, Governi che possono avere il tempo in cinque anni di portare avanti il proprio programma e che verranno giudicati alla fine della legislatura dagli elettori e quindi confermati o bocciati con l'elezione di una coalizione diversa rispetto a quella che ha appena governato. Questo è il modello dell'alternanza in cui noi crediamo e solo introducendo il premio di maggioranza in Costituzione ed evitando le contestazioni della Corte costituzionale alle leggi che sono state via via approvate si può trovare una soluzione. Il problema è chiaro, come abbiamo detto. La soluzione, secondo noi, principale è questa: il premio di maggioranza. ci si può dividere successivamente sulle modalità con cui assegnare il premio di maggioranza. C'è un bivio sostanziale: il premio di maggioranza può essere assegnato ad una pluralità grazie al consenso di un singolo, il *leader*, o l'indicazione del *Premier* può essere determinata grazie al premio di maggioranza assegnato ad una pluralità rappresentata dagli eletti di una coalizione che è risultata la più votata alle elezioni. Da una parte si premia, come modello per assegnare il premio di maggioranza, l'omogeneità della coalizione e il programma presentato agli elettori, dall'altra si premiano invece il carisma e le qualità del *leader* che rappresenta la coalizione. Sono tutti e due modelli legittimi e ognuno di noi può avere la preferenza per uno o l'altro di questi modelli. Una cosa è certa: entrambi garantiscono governabilità, stabilità e finalmente un'azione di governo chiara agli occhi degli elettori, che è il requisito fondamentale per poter giudicare l'operato di una maggioranza di Governo, senza che le forze politiche possano rimpallarsi responsabilità a seconda delle composizioni dei Governi che si succedono in una stessa legislatura. Credo che un esempio del fatto che le cose non funzionano e che non possono andare avanti in questo modo lo abbiamo sotto gli occhi. Tutti noi dovremmo

ha portato avanti in modo efficace quella misura. Ricordiamo tutti le parole di Draghi nelle Aule parlamentari con cui aveva sempre condannato l'introduzione di quel modello che avrebbe creato enormi problemi ai conti pubblici. È evidente che una misura ha bisogno di tempo per evidenziare i propri punti di forza e le proprie carenze, ed è solo la legislatura che può dimostrare questa alternativa tra le due considerazioni. Signora Presidente, di fronte al bivio se lasciare le cose come stanno o approvare un modello di premierato per migliorare la situazione attuale, noi crediamo che la scelta sia obbligata, obbligata, perché il Paese non può continuare ad avere Governi instabili, non può aver continuare ad avere maggioranze instabili e cambi di casacca. Grazie al lavoro del ministro Casellati e della maggioranza che ha trovato una unità di intenti all'interno della Commissione (dove il confronto in realtà c'è stato ed è stato anche molto approfondito), attraverso questa riforma possiamo dire che verranno raggiunti degli obiettivi importanti. In definitiva diciamo sì al premio di maggioranza, sì al Governo di legislatura, sì alla stabilità dell'azione di Governo, sì alla democrazia dell'alternanza: questi sono valori in cui crediamo e sono pienamente inseriti all'interno di questa riforma

Signora Presidente, la presenza del Governo continua è sicuramente un segnale positivo di attenzione e di ascolto, e parto da qui per dire che quando ci si avvicina a una riforma così delicata, una riforma istituzionale che pone il tema di cambiare, di fatto, la forma di governo del nostro Paese, la forma di governo parlamentare, si dovrebbe si dovrebbe farlo con prudenza ed equilibrio, ben sapendo che, quando si tocca la Costituzione, la si tocca interpretando lo spirito dei tempi, non con la testa rivolta al passato. Oggi, quando noi andiamo a legiferare costituzionalmente, dobbiamo tenere presente la sfida che viene posta alle democrazie liberali, perché se la politica ha l'ambizione di guidare i processi di cambiamento e di accompagnarli, deve avere ben chiaro il contesto. Oggi noi affrontiamo una sfida senza precedenti rispetto a regimi autoritari che, rispetto al passato, sono riusciti a coniugarsi con sistemi di economia di mercato più o meno funzionanti, l'accusa rispetto alle democrazie liberali è che non c'è solo quel modello ad essere resiliente all'interno della sfida della competizione internazionale. internazionale. Noi invochiamo la difesa e la tutela delle democrazie liberali, ma non lo dobbiamo fare solo quando dobbiamo giustamente chiedere ai Paesi europei, agli Stati Uniti e ai *partner* internazionali di unirsi nell'affrontare l'aggressione russa. Lo dobbiamo fare anche quando in gioco ci sono i principi e i valori fondamentali scolpiti nelle nostre Costituzioni, ivi compreso uno dei principi cardine, nel solco del quale sono state costruite le nostre Istituzioni, cioè quello dell'equilibrio e della separazione dei poteri. Nel 1748 in «Lo spirito delle leggi», Montesquieu lo diceva chiaramente, quando scriveva che, affinché non si possa abusare del potere, occorre che il potere arresti il potere. Io parto da lì. Questa riforma garantisce l'equilibrio e la separazione dei poteri, perché la garantisce il presidenzialismo. Il presidenzialismo la garantisce. Noi non lo condividiamo e abbiamo anche spiegato perché. Lo hanno fatto molto bene soprattutto i senatori Giorgis e Parrini nelle Commissioni competenti, anche perché negli Stati Uniti c'è un Presidente fortissimo, con dei poteri ben definiti, ma un Congresso altrettanto forte che, quando vuole impedire al Presidente di far passare delle leggi, arriva fino allo *shutdown*: non si pagano, cioè, gli stipendi e le pensioni.

diretta del Presidente del Consiglio, per quel combinato disposto scellerato della previsione di una legge elettorale con premio di maggioranza. Lo strascico, con cui il Presidente del Consiglio eletto direttamente dal popolo si porterebbe tutti i parlamentari, schiaccia il legislativo sull'esecutivo, financo ad arrivare a toccare la previsione dei *quorum* di garanzia che, nel momento in cui si ha una maggioranza di quel genere, incide sulla scelta dei membri del CSM, incide sulla scelta dei membri della Corte costituzionale.

di essere messa in chiara difficoltà. Questo è uno dei punti fondamentali ed è un motivo per cui nessuna democrazia liberale ha mai adottato un sistema di elezione diretta del Presidente del Consiglio. Il rischio è questo: manca il rispetto della separazione dei poteri, manca l'equilibrio dei poteri. Perché, nel momento in cui si ha una legittimazione diversa nelle elezioni dei vertici, dei due Presidenti, il Presidente del Consiglio eletto dal popolo e, dall'altra parte, un Presidente della Repubblica eletto dal Parlamento, si ha una fonte di legittimazione diversa. E poiché la storia si incarica di richiamarci ai precedenti, a come, in quel passaggio del 2019, addirittura si arrivò a invocare l'*impeachment* del presidente Mattarella, perché si era osato dire che questi non poteva esprimere la valutazione su un Ministro che gli era stato proposto; figuriamoci davanti a una diversa legittimazione tra Presidente del Consiglio eletto con una forte legittimazione popolare ed invece un Presidente da Repubblica eletto dal Parlamento: a quel punto, il primo si sentirebbe unto del Signore, forte della volontà popolare prevaricante dei poteri scritti nella Costituzione, che rischiano di non essere rispettati. Questo è un rischio evidente e umilia il Parlamento. Quella sarebbe davvero l'emergenza da trattare. Tornerò fra poco sulle prerogative del Parlamento, che a quel punto verrebbero schiacciate per i motivi che dicevo prima e per il fatto di non affrontare le vere emergenze. L'abuso della decretazione di urgenza è una di queste insieme al fatto che, ormai, i disegni di legge parlamentare sono stati messi su una corsia secondaria.

noi non dobbiamo stare con la testa rivolta al passato, perché ogni fase politica, ogni epoca, ha un suo sistema. Oggi il mondo sta cambiando a velocità impressionante, con la globalizzazione che ha cambiato la competizione, con i conflitti identitari dovuti alla crescita dei flussi migratori, con la transizione ecologica digitale e società sempre più polarizzate. Davvero pensiamo di poter paragonare il 2024 alla fine degli anni Novanta, quando il mondo è cambiato? *(Applausi)*. È evidente che questi sono i tempi che ci è dato di vivere ogni fase politica richiede sistemi istituzionali resilienti e capaci di rispondere a quelle sfide. Oggi i territori sono in competizione fra loro per attrarre investimenti, turisti, risorse. Non c'è più l'ombrello dello Stato nazione; la complessità della *governance* per tenere insieme autonomie locali e Stati nazionali. L'Europa richiede presidenti garanti e arbitri e noi vogliamo tenerci un Presidente solo perché si chiama Sergio Mattarella (anche perché si chiama Sergio Mattarella, che ha dimostrato di avere grande equilibrio) *(Applausi)*. Abbiamo bisogno di una figura di garante della Costituzione e di arbitro, in cui si riconosca la maggior parte del corpo elettorale e dei cittadini, che sia altresì garante della coesione nazionale. Noi affronteremo fasi complicate e difficili con la transizione ecologica e digitale che non sarà un pranzo di gala. Avere un Presidente che ci tenga insieme, ricoprendo quel ruolo di arbitro e garante, è un valore che noi vogliamo tutelare.

Ministra delle riforme, noi siamo stati molto chiari. Ce ne dovete dare atto. Fin dal primo momento, abbiamo detto in maniera molto chiara che avevamo una linea rossa: no all'elezione diretta del Presidente della Repubblica, no all'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Siamo stati leali, chiari e trasparenti, ma allo stesso tempo abbiamo presentato le nostre proposte e abbiamo detto che sul tema dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio non avremmo fatto riduzione del danno, non ci saremmo piegati a negoziare, a portare a casa un emendamento. Come abbiamo detto fin dal principio, noi siamo disposti a ragionare sull'efficacia dell'azione di Governo, sulla stabilità degli Esecutivi e sul rafforzamento delle prerogative del Parlamento, che oggi è la vera emergenza. Ve lo vogliamo dire in maniera molto chiara e molto netta: fermate lo scambio fra autonomia differenziata e premierato e noi ci sediamo al tavolo un secondo dopo. *(Applausi).* Ci sediamo per parlare del modello che ha garantito stabilità ed efficacia del Governo in maniera senza eguali a livello continentale, quello tedesco. I numeri parlano chiaro: in Italia, 31 Presidenti del Consiglio, 68 Governi, 9 cancellieri, 24 Governi. Molto più del modello britannico, dove abbiamo visto, solo nell'ultima legislatura, avvicendarsi almeno tre *Premier* diversi. Il modello tedesco prevede nomina e revoca sfiducia costruttiva. Qualcuno dice che è stata utilizzata una sola volta. È chiaro che è stata utilizzata una sola volta perché ha funzionato come deterrente e ha garantito la stabilità di quei Governi. Ripartiamo da lì, poi discutiamo modello tedesco fino in fondo. Noi siamo disponibili a discutere di tutto se voi vi fermate e tornate al tavolo di discussione. Ricordo che dopo quell'incontro non abbiamo più avuto neanche risposta sui temi che abbiamo portato, sulla sfiducia costruttiva, sul voto con provvedimenti a data certa e su un ragionamento serio. Le democrazie liberali si reggono anche sulla qualità della nostra democrazia e sui partiti. Riguardo la riforma dell'articolo 49 della Costituzione e i partiti, siete o non siete d'accordo con l'idea di inserire regole trasparenti? Una democrazia funziona se ci sono partiti sani con regole trasparenti che sappiano scegliere la propria classe dirigente. Sono questi i temi su cui noi ci siamo: sfiducia costruttiva, nomina e revoca, Parlamento in seduta congiunta, innalzamento dei *quorum* di garanzia, capacità di superare le liste bloccate e far scegliere davvero i cittadini. Il messaggio infatti del "decidi tu" è un messaggio sottile

non ci rassegneremo e faremo una battaglia parlamentare fino in fondo per difendere i principi scolpiti nella nostra Costituzione e salvaguardare un equilibrio che i nostri Padri fondatori hanno voluto e che noi vogliamo conservare, proiettandoci verso il futuro.

anche quelli del MoVimento 5 Stelle, di cui purtroppo non abbiamo nessun esponente in Aula al momento, anzi no, ce ne sono due. *(Commenti).* Poco fa noi eravamo solo dieci e hanno detto che non c'era nessuno. Per carità, ciascuno ha i suoi impegni, può valere anche all'inverso. ho tratto innanzitutto una buona notizia dal complesso degli interventi dell'opposizione, perché la maggior parte di essi dicevano che questa riforma, alla quale sono evidentemente contrari, serve per dare maggiori poteri a Giorgia Meloni e all'attuale Governo. Governo. Siccome ovviamente questa riforma entrerà in vigore con le prossime elezioni, vuol dire che i colleghi dell'opposizione sono sicuri che vinceremo di nuovo noi.

potremmo continuare non soltanto fino al 2027, ma anche in seguito con il Governo che ha dato risultati già in questo primo anno e mezzo, nonostante la situazione estremamente difficile a livello internazionale e nonostante l'enorme peso economico costituito da colpi di genio come il superbonus e altri che peseranno

a meno che voi riteniate che abbiamo già vinto noi, potrebbe anche riguardare i vostri Governi, che potrebbero anch'essi avere una maggiore stabilità. Il senatore Alfieri, intervenuto poco fa, ha ricordato i numeri, ma da questi numeri poi bisogna trarre delle conseguenze. Se negli ultimi quarant'anni, nei quarant'anni precedenti l'inizio dell'attuale Governo, l'Italia ha avuto 28 Governi diversi, la Germania 12

è un'altra cosa.

dire che con questa riforma una maggioranza che potrebbe non aver ottenuto la maggioranza dei voti dai cittadini potrebbe - pensate un po' - avere la maggioranza alla Camera e al Senato, potrebbe - orrore, orrore - eleggere un Presidente della Repubblica che appartiene a quella maggioranza. È una cosa terribile agli occhi di chi preferisce invece stare al Governo senza vincere e avere sempre e avere sempre la garanzia che in qualche modo ci si aggiusta per restare al Governo e controllare ampie fette di potere.

non è il contenuto della riforma, ma chi la sta facendo. Se la fa il centrosinistra, va benissimo modificare 53 articoli, va benissimo approvare una legge elettorale che avrebbe alla maggioranza nell'unica Camera vera, perché il Senato sarebbe stata una sorta di dopolavoro per consiglieri regionali e sindaci;

Non ho visto segni di pentimento, nessuno ha detto che aveva sbagliato all'epoca. Non lo so, si vede che il processo è stato molto intimo e nessuno ne ha avuto notizia. Quanto poi alle leggi maggioritarie, ricordo che non ci sono solo quelle col premio di maggioranza, e che anche i collegi uninominali o la prevalenza di collegi uninominali hanno degli ampi effetti maggioritari. La legge che ha governato le elezioni dal 1994 al 2001

Romano Prodi, con la sua coalizione, con il 43,4 per cento dei voti. Anche all'epoca era un obbrobrio? Mi permetto di ricordare che quella legge si chiamava Mattarellum il nome suggerisce chi l'ha proposta. *(Applausi)*. Allora, se le leggi con effetti maggioritari sono un obbrobrio per la democrazia (cosa che io non credo), allora questo è uno di quei famosi attacchi alla figura alla figura istituzionale che tutti rispettiamo e che dunque non ci sogneremmo di attaccare; tuttavia, certo che se si dice che si dà la maggioranza a chi non ha una maggioranza nell'elettorato, allora c'è un implicito attacco. Poi ho sentito parlare di Parlamento al guinzaglio, di parlamentari burattini e così via. Si dice questo perché, per far cadere il Presidente del Consiglio eletto, bisognerebbe sfiduciarlo e, di conseguenza, avere l'alta probabilità (in alcuni casi la certezza, su scelta del Presidente del Consiglio sfiduciato) di andare alle elezioni. che nella storia della nostra Repubblica questo è successo molte volte: nel 1979, nel 1983, nel 1976, nel 1987, nel 1996, nel 2008, nel 2013 e nel 2022. Il Parlamento non diede la maggioranza al Governo al quale avrebbe potuto darla, ben sapendo che si sarebbe andati alle elezioni. Pertanto il Parlamento non è servo del Governo per il fatto che se cade il Governo si va alle elezioni; il Parlamento ha avuto e ha la sua autonomia ed ha il potere (anche con questa riforma non cambierebbe nulla rispetto a tutti i numerosi casi che ho citato) di cambiare Governo, di togliergli la fiducia e

ha aumentato di molto il debito pubblico e ha mortificato l'economia italiana, rendendola preda di varie operazioni finanziarie internazionali. C'è un altro aspetto che vorrei sottolineare. Il presidente Monti ha detto che non saranno più possibili Governi di unità nazionale. Non è vero, perché se c'è un'emergenza, nulla vieta di avere unità nazionale come succede praticamente in tutte le altre democrazie, se c'è il momento in cui bisogna stringersi a coorte.

dei tecnici, persone non elette da nessuno, non è obbligatorio e in democrazia dovrebbe essere veramente una ipotesi da escludere, anche se è successo e noi lo rispettiamo. Naturalmente era tutto fatto nel rispetto della Costituzione, con un ultimo elemento. Si evocano pericoli per la democrazia e le dittature del secolo scorso, naturalmente non quelle comuniste, perché, come ci insegna la senatrice Maiorino, di quello che succede all'estero non ci interessa niente. Il presidente Pera ha dato una lezione su come funziona la più antica democrazia del mondo, ma quello non c'entra perché avevano il re, gli hanno tagliato la testa; noi non abbiamo tagliato la testa al re, dunque non possiamo fare paragoni e dunque cade anche la questione di dire che altrove non c'è l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. nel 1921 ci furono le elezioni parlamentari in Italia e furono elezioni regolari; i deputati di Benito Mussolini furono eletti nella misura del 6,5 non mi sembra una misura sufficiente per vincere le elezioni presidenziali. Se ci fosse stata l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, non mi pare che Mussolini sarebbe potuto diventare Presidente del Consiglio. Lo divenne con meccanismi che per l'appunto hanno consentito al Capo dello Stato di fare scelte sue, valutando le opportunità e magari facendo un Governo che poteva essere visto come di salvezza nazionale. *(Proteste.

erano quelli (mica perché aveva preso il 90 per cento dei voti e poi ha deciso di prendere solo quelli). Ricordo anche che in Germania il partito nazionalsocialista arrivò al potere

Ricordo che alle elezioni presidenziali, quando i tedeschi scelsero chi doveva essere il Presidente con voto diretto (e il cancelliere non era scelto con voto diretto), Hitler fu battuto da Hindenburg 49 a 30 nel primo turno e 53 a 36 nel secondo turno. Non dite pertanto che il pericolo dell'elezione diretta è quello, perché mi sembra che con l'elezione diretta i due più celebri dittatori del secolo scorso

ci sia una maggiore garanzia per i cittadini e del rispetto dei diritti costituzionali, che sono sacri e non vanno toccati neppure quando ci sono le emergenze.

Signor Presidente, cari colleghi, ho ascoltato con attenzione gli oltre settanta interventi delle opposizioni e devo dire che mi sono sembrati sostanzialmente tutti uguali, ripetitivi sempre degli stessi argomenti e delle stesse obiezioni, al netto ovviamente, caro Presidente, degli insulti,

le riforme si fanno tutti insieme, ci hanno ammonito i colleghi dell'opposizione. Giusto: peccato che quando noi li esortavano in questo senso, ad esempio in occasione della riforma del Titolo V della Costituzione, i colleghi che oggi ci esortano a fare le riforme tutti insieme ci ricordavano che esiste l'articolo 138 della Costituzione. Colleghi, ma è stato abrogato l'articolo 138 della Costituzione dal 2001 a oggi? A sentire voi, sembrerebbe di sì. O è stato abrogato dopo la riforma Boschi-Renzi, altra occasione nella quale l'articolo 138 della Costituzione ve lo siete scordato? I Padri costituenti non hanno scritto anche l'articolo 138 della Costituzione, per caso? E ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, non sarà alla fine il popolo a decidere con un suo voto sovrano se questa riforma riceve il consenso del corpo elettorale oppure no? Non si chiama democrazia? O non avete fiducia nel popolo italiano? È una domanda legittima.

osservazioni. Non è così, perché le audizioni che si sono tenute in Commissione affari costituzionali ci hanno consentito di migliorare sensibilmente questo testo. È stato inserito il limite ai mandati ed è stato tolto un premio troppo rigido del 55 per cento determinato in Costituzione. È stato poi risolto un problema che tantissimi costituzionalisti e anche molti colleghi dell'opposizione avevano sollevato: così come era scritta la norma inizialmente, si rischiava il paradosso di un secondo *Premier* che contasse più del primo. Leggendo l'emendamento che abbiamo approvato in Commissione, scoprirete che non è più così: qualsiasi sia la causa della crisi che si dovesse determinare, sarà sempre il *Premier* eletto ad avere l'ultima parola. Quindi, credo che invece abbiamo ascoltato. Cos'è, colleghi, che non potevamo ascoltare? Non potevamo ascoltare una minoranza che pretendeva di avere il potere di veto sulla maggioranza. Questo è stato l'atteggiamento delle opposizioni. Quando in Commissione viene il senatore Alfieri, responsabile delle riforme per il Partito Democratico, e ci dice che, fino a quando noi manterremo l'elezione diretta del *Premier*, non saranno disposti a collaborare e a contribuire contribuire a migliorare il testo, perché deve essere soltanto cestinato, è chiaro che non ci lasciavate altra scelta. Vi do una notizia, cari colleghi: il disegno di legge si intitola elezione diretta del *Premier*. Se uno non vuole discutere dell'elezione diretta del *Premier*, è chiaro che non c'è più nulla di cui discutere. E lo avete dimostrato, con decine e decine, centinaia di interventi ripetitivi all'ossessione sempre degli stessi argomenti, con 2.600 emendamenti in Commissione, con 3.000 e oltre emendamenti oggi presentati in Aula. Sono legittimi, siamo in democrazia, ci sono i Regolamenti parlamentari. Ripeto ma non potete adesso lamentare il fatto che, a fronte di questo vostro atteggiamento pregiudizialmente avverso e assolutamente ostruzionistico, la maggioranza eserciti la prerogativa che

fa la maggioranza. Non potete risentirvi di una mancanza di dialogo che voi per primi avete solennemente annunciato di rifiutare. Seconda obiezione: dite che questa riforma indebolisce il Parlamento, perché il Parlamento verrebbe eletto a strascico del *Premier*. Sbagliato.

questa riforma avrà un effetto bipolarizzante del sistema: ci saranno due coalizioni che, se vorranno competere, dovranno tendere a comprendere ben più del 40 per cento, non soltanto in caso di vittoria, ma anche in caso di sconfitta. Ci avviciniamo cioè, finalmente, a quel bipolarismo compiuto e a quella democrazia dell'alternanza che - a mio modesto parere e a parere di tutto il centrodestra - è l'unica vera forma di democrazia compiuta. Ma c'è di più: cari colleghi, vi siete accorti che in realtà oggi il Parlamento è deciso da una manciata di persone? Vi siete accorti che voi siete stati tutti eletti con le liste bloccate? Sapete chi scrive le liste bloccate? Le scrivono i *leader* dei partiti. Ma, fino a quando le liste bloccate le scrivono i *leader* dei vostri partiti - chissà perché - non vi scandalizzate del

L'Italicum lo avete votato voi. Il Rosatellum l'ha votato il PD, che oggi si lamenta del sistema elettorale che prevedrà un premio di maggioranza per il *Premier* eletto e si scandalizza, anche se abbiamo annunciato che introdurremo le preferenze. Per cui sarà certamente molto meno a strascico o per trascinamento di quanto sia stato questo e il precedente Parlamento, tanto più che - come sapete - col Rosatellum anche i collegi uninominali sono uninominali per modo di dire, perché non c'è modo di votare un candidato diverso Il partito votato trascina automaticamente il voto anche sul candidato dell'uninominale. Qualcuno ha detto che con questa legge ci può essere un sistema per cui, con il 25 per cento dei voti, si prende la maggioranza assoluta dei seggi: sbagliato, cari colleghi; quello era l'Italicum, dove era previsto un ballottaggio tra liste, per cui una lista, che andava al ballottaggio con il 55 per cento, si poteva prendere il 55 per cento dei seggi. Quel sistema l'avevate scritto voi. Non c'era un problema di democrazia con l'Italicum, cari colleghi? C'è adesso il problema di democrazia? altro argomento è che vengono indeboliti i poteri del Presidente della Repubblica:

con questa riforma viene enfatizzato, non viene mortificato. Con questa riforma viene enfatizzato il ruolo di arbitro del Presidente della Repubblica, di garante dell'unità nazionale di custode della Costituzione. Il Presidente della Repubblica continuerà a presiedere il Consiglio superiore della magistratura; continuerà a presiedere il Consiglio supremo di difesa; continuerà a nominare i cinque giudici della Corte costituzionale, anche grazie a un emendamento del presidente Pera che ha chiarito che quell'atto non è soggetto a controfirma; continuerà a inviare i messaggi alle Camere; continuerà a respingere i progetti di legge del Governo manifestamente incostituzionali e continuerà a promulgare le leggi con la possibilità di rifiutare la firma. Questi sono i ruoli di garanzia e di custode della Costituzione, che non solo il Presidente della Repubblica mantiene, ma che vengono anche ulteriormente valorizzati. Tra l'altro, vi segnalo che, grazie a un emendamento del Governo, il Presidente della Repubblica non soltanto nominerà i Ministri, ma li potrà anche revocare e, quindi, è un potere in più. il Presidente della Repubblica non nominerà più i senatori a vita. Pensate un po', cari colleghi: il centrodestra si ritrova nella stessa identica posizione in cui si trovò il Partito Comunista Italiano in sede di Costituente, quando votò contro la norma che riguardava la nomina dei senatori a vita, perché - pensate un po' riteneva che in Parlamento, in una democrazia, ci si venga solo su mandato del popolo sovrano. Siamo d'accordo su questo principio sancito in Costituente dal Partito Comunista, mentre voi ritenete che, seppur soltanto in numero limitato, in Parlamento ci si possa venire anche non su mandato del corpo elettorale. Eppure, paradossalmente, saremmo noi gli antidemocratici e gli autoritari. Va bene, ne prendiamo atto. A parte questo limitato caso, i poteri del Presidente della Repubblica restano gli stessi. Certo, non potrà più svolgere quel ruolo di supplenza che ha svolto in determinati momenti di crisi del sistema, quando il sistema non è stato all'altezza del compito ed ha costretto il Presidente della Repubblica,

semplice: con l'elezione diretta non ce ne sarà più bisogno, poiché risolviamo a monte i problemi creati dalla instabilità politica cronica del nostro sistema. Colleghi, l'instabilità non è soltanto un *vulnus* per la democrazia ma - come hanno dimostrato molti studi - è anche un vulnus per l'economia, se è vero come è vero che l'instabilità

ma la legittimazione in una Repubblica democratica non viene dalla Costituzione? E la Costituzione non legittima ugualmente il *Premier* eletto il Presidente della Repubblica eletto dal Parlamento? La legittimazione risiede nella Costituzione per l'uno e risiede nella Costituzione per l'altro. Certo, se vogliamo valorizzare il ruolo di arbitro *super partes* del Presidente della Repubblica, dobbiamo anche accettare il fatto che debba essere eletto con un sistema che ne valorizzi il ruolo di unità, non certo il ruolo divisivo che esprime un capo della maggioranza, di qualsiasi maggioranza, nel momento in cui viene eletto direttamente.

regolarmente, ogniqualvolta il mio interlocutore si è trovato in difficoltà e non ha avuto più argomenti, ha tirato fuori il fascismo. *(Applausi)*. Se il fascismo come arma dialettica non esistesse, la dovreste inventare.

vi invito a fare una ricerca storica, visto che qualcuno ha citato le ricerche storiche. Andate a studiarvi chi era Stanis Ruinas. *(Applausi)*. C'è un bellissimo libro di Paolo Buchignani e si intitola «Fascisti rossi». Andate a studiare i rapporti del fascista di sinistra, Stanis Ruinas, aderente e militante della Repubblica Sociale Italiana, negli anni 1945 e seguenti, con Palmiro Togliatti e con Botteghe Oscure, per portare una quota importante di fascisti repubblicani della RSI

chi erano i fascisti in camicia rossa. La storia o la studiate tutta o la lasciate perdere. *(Applausi)*. Parliamo del futuro. Parliamo di come migliorare le nostre istituzioni. Parliamo della nostra Costituzione, che è certamente la più bella del mondo, che certamente tutti noi sottoscriviamo dalla prima all'ultima parola, comprese le disposizioni transitorie finali, ma parliamo del futuro. È questo, infatti, che interessa agli italiani.

Signor Presidente, vorrei ringraziare il relatore, senatore Balboni, per l'accorto e paziente lavoro degli ultimi mesi, e tutti i senatori, che ho ascoltato con attenzione e interesse, intervenuti qui oggi nel dibattito sulla riforma costituzionale; una riforma che ho affrontato muovendo da una ricognizione oggettiva e non ideologica dei problemi che affliggono la forma di governo. In via preliminare, sento davvero il dovere di rispondere alla critica di non aver cercato fino in fondo il confronto con le minoranze sui contenuti della riforma; una critica che trovo francamente ingenerosa, alla luce dei numerosi incontri che ho personalmente tenuto con tutte le forze politiche nei mesi che hanno preceduto preceduto la formalizzazione del disegno di legge governativo. In quelle occasioni, tutti i rappresentanti delle forze politiche di opposizione hanno chiesto di non perseguire la strada di una riforma in senso presidenziale, un mutamento che era stato ritenuto troppo radicale e che avrebbe messo a repentaglio la funzione di garanzia e terzietà del Capo dello Stato. Da molti dei partiti di opposizione è emersa la richiesta di aderire, piuttosto, alla soluzione del rafforzamento della figura del Presidente del Consiglio dei ministri. Nonostante il nostro programma prevedesse l'opzione presidenziale, ho preso atto di queste sollecitazioni e ho orientato la proposta del Governo in questa direzione. Allo stesso modo, il confronto è proseguito in Commissione, dove sono stati accolti numerosi suggerimenti, anche provenienti dalle opposizioni. A fronte di questi fatti, semplici e conclamati, sentirsi accusati oggi, senatori Parrini e Giorgis, di aver rifiutato in maniera aprioristica il confronto lascia davvero stupefatti. Di converso, le dichiarazioni plurime delle opposizioni dall'inizio dell'esame del testo di riforma sono state sempre inconciliabili con uno spirito costruttivo: il testo inemendabile; siamo contrari su tutto; non accettiamo l'elezione diretta; la presentazione di 2.600 emendamenti in Commissione e più di 3.000 emendamenti in Aula; nessuna proposta alternativa. Sono circostanze che si commentano da sole. Sono stati alzati muri ideologici, per di più contraddittori. Il Partito Democratico, che si è opposto al premierato per una presunta diminuzione dei poteri del Capo dello Stato, ha poi fatto accenno al modello tedesco del cancellierato, che riduce il suo ruolo ad un esercizio meramente notarile. Il MoVimento 5 Stelle, che ha predicato il valore imprescindibile della consultazione popolare per dare risposte su ogni tema, si è opposto poi al diritto fondamentale dei cittadini di scegliere il proprio *Premier*. Si è sostituita la mancanza di argomentazioni giuridiche con *slogan* del tipo "Barattellum tra riforma costituzionale e autonomia differenziata", fingendo di dimenticare che entrambe le riforme fanno parte del nostro programma elettorale. Fatta questa premessa, la nostra storia istituzionale ci restituisce numeri impietosi. In settantasei anni ci sono stati 68 Governi, con la durata media di La riforma approdata in quest'Aula non è quella del e per il centrodestra: è una riforma per l'Italia. come avete detto ripetutamente - che il nostro tentativo è inutile perché tanto i cittadini la bocceranno al *referendum* e che stiamo lavorando oggi solo per piantare bandierine e fare propaganda elettorale in vista delle elezioni europee, vuol dire che state riconoscendo direttamente che la nostra riforma costituzionale risponde alle richieste e agli interessi dei cittadini elettori. allora sulla strada giusta. È una riforma per l'Italia, che intende dare risposte a quelli che tutti - dico tutti tutti - hanno avvertito come la zavorra più pesante per il nostro sistema istituzionale: la mancanza di stabilità degli Esecutivi e la mancanza di continuità di un indirizzo politico. Già i Padri costituenti ne ebbero piena consapevolezza ed essa si tradusse nel famoso ordine del giorno Perassi, che restò però inattuato. Da qui i limiti e le degenerazioni dell'odierno parlamentarismo, dimostrati da quarant'anni di tentativi, da destra e da sinistra, di modificare la forma di governo. Da qui l'epiteto di malato d'Europa, affibbiato all'Italia dal giornale «The Economist», per la perenne instabilità dei Governi, per l'alta frammentazione dei partiti, per il trasformismo parlamentare, per la costante supplenza del Capo dello Stato e per il ricorso ai Governi Una delle cause dell'instabilità dei Governi è stata la fragilità dei poteri di direzione politica del Presidente del Consiglio. Questa riforma ne rafforza il ruolo, dotandolo di una robusta legittimazione politica che deriva dall'elezione diretta. Avete criticato la scelta di far eleggere il Presidente del Consiglio dal popolo perché comporterebbe il rischio di una deriva autoritaria, la lacerazione del tessuto costituzionale e la rottura dell'ordine repubblicano; il tutto aggravato dalla crisi dei partiti. Non la pensava così Cesare Salvi, esponente del Partito Democratico, che osservava come l'elezione diretta non potesse dar luogo a degenerazioni plebiscitarie o a pericoli per la tenuta democratica del sistema istituzionale; così come la legittimazione popolare - sosteneva sempre Salvi - era idonea a sollecitare la rivitalizzazione dei partiti. Non la pensavano così neppure i senatori del Partito Democratico Parrini e Ceccanti, che presentarono due disegni di legge nella legislatura del 2018 - quindi ieri - sull'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Del resto, non potrebbe essere altrimenti. Con questa riforma, infatti, finalmente la Costituzione si riconcilia con il principio di sovranità popolare, perché affida agli elettori la scelta non solo dei loro rappresentanti in Parlamento, ma anche di chi li governerà. Mi potete spiegare perché i cittadini non devono sapere e devono essere tenuti all'oscuro di chi li governerà? Il voto è la prima e la più alta forma di partecipazione alla vita democratica e il disallineamento tra voto degli elettori e guida del Governo è una delle cause della disaffezione politica che ha portato a un galoppante e preoccupante astensionismo dalle urne elettorali. Noi non ci rassegniamo a considerare i cittadini figli di un Dio minore, perché siamo convinti che il popolo non abbia bisogno di un costante tutoraggio, come se fosse un bambino mai cresciuto. Siamo convinti che i cittadini debbano tornare a esercitare il potere di scelta del proprio Governo senza alcun timore di tiranni o di Cesari che sono consegnati per sempre a una storia che nessuno - dico nessuno - vuol far tornare e che non tornerà mai. Ritenete davvero che si preservi la pienezza del dibattito democratico e del pluralismo, senatori Giorgis e Camusso, con l'abilità nel giocare l'eterno gioco dell'intrigo, il gioco del ribaltone, dei Governi tecnici? Ritenete che possa perpetrarsi ciò che è accaduto specialmente negli ultimi dieci anni e particolarmente nella scorsa legislatura, dove maggioranza e opposizione, anziché presentarsi come due schieramenti chiaramente contrapposti, hanno finito per porsi come due vasi comunicanti alla faccia della responsabilità politica nei confronti degli elettori? Se questa è la vostra proposta, la risposta che diamo attraverso la riforma è un netto no, perché il voto popolare è il faro che deve orientare la dinamica democratica, che non può e non deve risolversi in una delega in bianco consegnata al Parlamento. che questo modello di premierato sarebbe estraneo alla cultura costituzionale e sarebbe senza precedenti a livello comparato se si esclude l'esperienza israeliana. Non è così: la scelta di eleggere il Presidente del Consiglio non è un fiore spuntato nel deserto, un'innovazione incompatibile con la nostra storia repubblicana. La prospettò in seno all'Assemblea costituente Costantino Mortati, uno dei più autorevoli costituzionalisti del Novecento, protagonista assoluto del dibattito sulla forma di governo, e la difese con forza Augusto Barbera, oggi Presidente della Corte costituzionale. Non c'è dubbio che il disegno di legge costituzionale abbia un suo tratto di originalità ed è per questo che ho più volte parlato di un premierato all'italiana. La forma di governo - come dicono insigni costituzionalisti - deve essere come un vestito che va adattato al nostro corpo sociale, un modello italiano e, quindi, più vicino alla sensibilità del nostro Paese. Ma mi chiedo e vi chiedo perché avete paura di una novità. Non hanno avuto paura i francesi con il semipresidenzialismo, modello oggi diffuso ma anch'esso completamente inedito - come è stato detto in quest'Aula più volte - circondato da un vasto scetticismo quando fu introdotto nella Costituzione francese della Quinta Repubblica. I 12 Stati europei che vi fanno riferimento non lo hanno adottato *tout-court*, ma lo hanno applicato alle proprie esigenze economiche, politiche e sociali in un diverso equilibrio di pesi e contrappesi tra poteri del Capo dello Stato e poteri del Presidente del Consiglio. Anche gli Stati Uniti e la Germania hanno inventato, rispettivamente, la forma costituzionale del presidenzialismo e del cancellierato, non senza preoccupazioni, non senza critiche. Non vedo, quindi, alcun problema nel fatto che l'attuale progetto di riforma sia un *unicum* e che l'unica forma ad esso assimilabile sia quella sperimentata in Israele. Il modello israeliano ha fallito perché è mancato il collegamento tra elezione popolare del *Premier* e garanzia di una maggioranza di sostegno al Governo, che è invece il tratto qualificante del disegno di legge che oggi stiamo esaminando. Avete criticato la riforma accostando la figura del Presidente del Consiglio eletto all'immagine di un *leader* solitario al comando, usando espressioni colorite come capocrazia, autocrazia elettiva e simili, che mi appaiono più adatte a uno *slogan* che a un punto di vista basato su argomenti giuridici. La conseguenza sarebbe quella di un Parlamento svilito, condannato ad essere piegato alla volontà del *Premier*, con parlamentari ridotti ad un'adunanza di militanti obbedienti e diligenti. A sostegno dell'assunto di un Presidente del Consiglio eletto come una sorta di asso pigliatutto, la cara amica senatrice Segre fa riferimento alla legge Acerbo del 1923, che prevedeva l'attribuzione dei due terzi alla lista che avesse superato il 25 per cento dei voti validi. Ma chi si è mai sognato di scrivere una legge di questo tipo? Nella riforma si fa riferimento a un premio di maggioranza legato al principio di rappresentatività - come è emerso nel dibattito in Commissione - non ho mai ipotizzato una soglia inferiore al 40 per cento, in sintonia con la giurisprudenza costituzionale. Non ci sarà neppure un'elezione a strascico, come piace raccontare a vari senatori: le elezioni dei dei due organi, Parlamento e Presidente del Consiglio, sono contestuali; le coalizioni proporranno agli elettori un programma di Governo ed un *leader* e liste di parlamentari. Ed è su questo pacchetto di di idee e di rappresentanti che gli elettori si pronunceranno, facendo emergere dal voto un chiaro indirizzo per la legislatura. Il cantiere della legge elettorale si aprirà - come ho già detto - dopo l'approvazione in prima lettura, con l'auspicio di una maggiore fortuna nella collaborazione con le forze di opposizione. L'elezione diretta del *Premier* è quella più in armonia con i poteri del Parlamento, perché attiene alla responsabilità politica. Il *Premier* risponde al Parlamento, sottoponendosi ai suoi poteri di controllo, fino alla rimozione da parte del Parlamento stesso; è vincolato agli indirizzi e alle risoluzioni del Parlamento; risponde meglio alle domande dei cittadini di eleggere il Governo. Sono parole non mie, ma dell'attuale presidente della Corte costituzionale, professor Augusto Barbera, che attribuisce al Parlamento un ruolo centrale, perché il Presidente del Consiglio può restare in carica per l'intera legislatura solo ed esclusivamente se gode del consenso del suo partito prima di tutto e degli altri partiti della maggioranza. Il Parlamento come acutamente osserva la senatrice Musolino - ha quindi il potere politicamente più rilevante e significativo, che è quello di dare e revocare la fiducia e, quindi, di fare e di disfare il Governo, oltre che la possibilità di rendere difficile al *Premier* l'attuazione del programma per la quale si è assunto la responsabilità davanti ai cittadini. Avete parlato di ricatto del Presidente del Consiglio, che terrebbe i parlamentari al guinzaglio in condizioni di subalternità. Mi rifiuto di pensare che questa critica sottintenda l'idea distorta di una politica politicante, dove i parlamentari eletti sarebbero costretti ad accettare tutto per mantenere la propria sedia, pur di non andare a casa. È un pensiero che respingo con forza, perché è uno schiaffo alla dignità personale e istituzionale di chi svolge un ruolo nel segno di un servizio alla comunità e non per interessi personali. Non mi difetta l'attenzione per la difesa delle prerogative di queste Aule parlamentari. La crisi del parlamentarismo non comincia con questa legislatura e non può essere imputata a questa riforma. È una crisi crisi che affonda le radici in problemi risalenti, cui hanno contribuito tutte le forze politiche che si sono succedute alla maggioranza negli ultimi anni. Mi è chiaro che in una Repubblica parlamentare come la nostra arginare la marginalizzazione del potere legislativo necessario, lasciando all'autonomia e all'autodeterminazione delle Camere la modifica stringente dei Regolamenti. È avvilente poi continuare ad ascoltare la stanca litania secondo la quale la riforma mortificherebbe la figura del Capo dello Stato. Alla base di questa critica c'è un profondo fraintendimento, che riguarda il ruolo dei due Presidenti della Repubblica e del Consiglio, che si muovono su due piani diversi e non sovrapponibili nell'assetto costituzionale. Il Presidente della Repubblica ha poteri di garanzia dei valori costituzionali e di rappresentanza dell'unità nazionale. La sua neutralità e la sua autorevolezza derivano dal fatto di non essere parte, ma di attingere la sua legittimazione dai valori della Costituzione. Le sue prerogative non sono state toccate, anzi, si sono aggiunti alla nomina anche la revoca dei Ministri e il potere solitario di firmare atti importanti che, nell'attuale sistema, condivideva con il Governo. Il Presidente del Consiglio ha invece poteri di indirizzo politico. Certo, la riforma limita le occasioni in cui lo Stato dello Stato - come ha osservato il professor Cassese - è costretto a dilatare la fisarmonica dei suoi poteri, come accadeva finora ogniqualvolta il sistema parlamentare andava in crisi. Io per prima riconosco i molti meriti dei nostri Presidenti della Repubblica nel gestire con sapienza fasi critiche del nostro sistema politico. Il nostro compito è però evitare - come ricordava il presidente Napolitano che quei momenti critici si ripetano. Ed è per questo che la riforma introduce per la prima volta un'articolata regolamentazione di tutte le crisi di Governo, disciplinando la responsabilità di fronteggiare le varie tensioni. E lo si deve fare proprio per salvaguardare l'autorevolezza del Capo dello Stato e metterlo al riparo dalle contingenze del Governo e dell'agone politico. È stato evocato anche il rischio che il premio di maggioranza possa implicare una sorta di cattura degli organi di garanzia. È falso e fuorviante: la Costituzione già richiede maggioranze qualificate per l'elezione tanto dei componenti laici del Consiglio superiore della magistratura quanto dei giudici della Corte costituzionale di elezione parlamentare, maggioranze qualificate che superano il perimetro delle maggioranze politiche anche in presenza di una maggioranza parlamentare supportata da un premio. Quanto al *quorum* per l'elezione del Presidente della Repubblica, tutti desideriamo garantire che sia scelto in base al più ampio consenso possibile. L'emendamento accolto in Commissione che prolunga al sesto scrutinio l'applicazione della maggioranza qualificata dei due terzi manifesta proprio l'obiettivo di promuovere logiche di dialogo e di condivisione nella selezione del Capo dello Stato. Avete detto che la riforma costituzionale serve non all'Italia, ma a distrarre l'attenzione dei cittadini dai tanti problemi che affliggono la nostra comunità. Io credo che tale affermazione sia grave e anche pericolosa: questo non è un dibattito filosofico ridotto a un'astratta contrapposizione dialettica, ma è una riforma su un tema che

dipendono la possibilità di fare impresa, la crescita economica, la fiducia dei mercati, la capacità di uno sguardo lungo verso il futuro,

se cambiano continuamente le regole del gioco. L'instabilità è costata, negli ultimi dieci anni, 240 miliardi di euro di interessi sul debito pubblico *(Commenti)*, una cifra superiore all'intero ammontare del PNRR. Sono denari, tanti, sottratti alle tasche degli italiani. Sono denari sottratti all'occupazione, sono denari sottratti agli investimenti. Questo è uno dei significati più profondi della riforma istituzionale. In conclusione, la riforma di cui discutiamo consolida la nostra democrazia, garantendo la stabilità delle istituzioni e rivitalizzando la dialettica politica e la rappresentatività degli organi costituzionali. riavvicinerà l'Italia alle grandi democrazie europee, nelle quali le istituzioni di governo ricevono dal corpo elettorale una legittimazione di indirizzo per la sua azione nel corso della legislatura, per poi sottoporre la valutazione del proprio operato nuovamente al corpo elettorale al termine della legislatura. Tutto ciò senza intaccare le prerogative del Parlamento di legiferare, controllare e correggere quotidianamente l'indirizzo politico del Governo, né la potestà del Capo dello Stato di esercitare i propri poteri di controllo e di garanzia dell'azione di Governo, né ancora la potestà della Corte costituzionale di cassare le leggi

L'Italia si avvia dunque a divenire una democrazia efficiente e di indirizzo, presidiata da solide garanzie costituzionali. È ciò che i cittadini chiedono da molti anni ed è questo il momento di realizzarlo. La ringrazio per il suo intervento molto chiaro.

erano anni, molti anni, che non si sentivano in quest'Aula parole di tanta demagogia qualunquista e antiparlamentare. Però è questo lo spirito del tempo, lo sappiamo, ed è anche lo spirito che anima questo Governo e parte significativa della maggioranza che lo sostiene. Voglio però prendere sul serio le considerazioni di chi, senza cedere all'antiparlamentarismo, pur essendo parlamentare, e senza cedere al qualunquismo, pur avendo responsabilità di governo, è entrato nel merito e ha suggerito di fermarsi di fermarsi e di affrontare questioni che sono rimaste aperte e che è molto difficile immaginare possano trovare soluzione nella legge ordinaria. È emerso in Commissione - lo sanno i colleghi della Commissione - ed è emerso in questa Aula, durante la discussione generale, come i molti cittadini italiani che risiedono in un Paese estero, e che magari non hanno mai vissuto neanche una giornata della loro vita in Italia, crescano continuamente e possano diventare determinanti per l'elezione

contraddice in maniera evidente il principio di democraticità. Il paradosso consiste nello scarto sempre più significativo tra coloro che sono sottoposti all'indirizzo politico che i nostri organi costituzionali definiscono e coloro che possono partecipare alla determinazione dello stesso indirizzo politico e delle stesse leggi. Uno dei profili essenziali del principio democratico, infatti, è quello di fare in modo che tutti possano concorrere a determinare le leggi a cui poi sono sottoposti. Noi invece ci troviamo in una curiosa situazione, in cui cresce il numero di coloro che non sono sottoposti alla nostra legge, perché non vivono in Italia e non hanno mai vissuto in Italia, e al tempo stesso cresce il numero di coloro che stabilmente vivono in Italia, lavorano e costruiscono legami, ma che, non potendo diventare cittadini, non hanno l'esercizio del diritto di voto. Insomma, noi siamo un Paese che vede ogni giorno aumentare questa forbice tra chi può eleggere i nostri organi e così, in qualche misura, concorrere a determinare l'indirizzo politico, e chi è sottoposto all'indirizzo all'indirizzo politico e alle leggi. È un problema molto serio che il presidente Pera ci ha ricordato in quest'ultima giornata, sollecitando il Governo e la maggioranza ad affrontarlo e soprattutto ad affrontarlo in maniera seria, cosa che, a Costituzione vigente e a riforma approvata in Commissione, non è possibile fare, perché nessuna legge ordinaria sarà in grado, da sola, di risolvere questa questione. Altro aspetto sul quale abbiamo cercato con serietà e con il massimo rigore possibile di argomentare è quello relativo al rapporto - che come abbiamo sentito adesso, secondo la Ministra, sarebbe del tutto risolto - tra garanzia del premio di maggioranza e garanzia del principio di rappresentatività. La riforma che avete scritto prevede che il Presidente del Consiglio eletto porti con sé una maggioranza parlamentare. Questo l'avete scritto in Costituzione; non avete voluto ascoltare le nostre perplessità e le critiche che hanno avanzato tutti coloro che abbiamo audito sull'impossibilità di tenere insieme la garanzia della maggioranza e la rappresentatività del Parlamento. Adesso ci venite a dire, come se fosse la cosa più ovvia del mondo, che questo premio non scatterà sempre, ma se non scatta sempre state già ipotizzando una palese violazione della riforma costituzionale che avete voi stessi scritto. Allora, forse un po' più di fiducia nel Parlamento, un po' più di fiducia nell'argomentazione, un po' più di umiltà nel rispondere alle critiche e alle obiezioni che sono state sollevate consentirebbe a tutti noi di fare un migliore servizio al Paese.

anche perché i comizi li avete fatti, avete replicato parlando ai vostri possibili elettori. Adesso il comizio è stato fatto,

la trattazione e la discussione sugli emendamenti a dopo le elezioni, sperando che ci sia un atteggiamento un po' più costruttivo e un po' più cooperativo da parte della maggioranza.

Devo dire che le due obiezioni che ha posto adesso il senatore Giorgis mi sembrerebbero, francamente, già di per sé largamente sufficienti per fermare questa discussione adesso. I due nodi posti non hanno avuto risposte e mi dispiace doverlo dire al presidente Balboni, che sa che ho apprezzato anche il lavoro fatto in Commissione, e alla ministra Casellati. C'è poco da discutere. Due obiezioni serissime sono state poste adesso dal senatore Giorgis. La prima è quella che riguarda l'incrocio tra premio di maggioranza e rappresentatività (chiamiamolo così); la seconda è la questione gigantesca degli italiani all'estero. Con tutto il rispetto per gli italiani all'estero, è davvero incredibile pensare di poter eleggere il Presidente del Consiglio con un voto così preponderante che accade fuori dai confini nazionali, per di più purtroppo un voto che spesso avviene con modalità anche opache, come ben sappiamo e come è stato riconosciuto mille volte. Trovo davvero incredibile che, dinanzi a queste due obiezioni così circoscritte, si faccia finta di nulla e si rimandi alla legge elettorale, che peraltro non conosciamo. Questa è un'altra cosa che considero molto grave: il fatto di arrivare in prima lettura

dalle senatrici e dai senatori dell'opposizione. Non è stata detta - mi dispiace dirlo anche in questo caso - nemmeno una parola sul tema di fondo che è stato sollevato, cioè sul rischio reale che venga messo in discussione l'equilibrio dei poteri. Soprattutto, trovo davvero incredibile che si continui a dire, come se fosse un disco rotto, una cosa negata nell'evidenza da questa riforma che proponete: come fate davvero a sostenere che non sono toccate le prerogative del Capo dello Stato, quando perlomeno su due questioni gigantesche *(Applausi)*, la formazione del Governo e lo scioglimento delle Camere, che sono due tra i principali poteri che la Costituzione attribuisce al Capo dello Stato, si cerca invece una strada che stravolge questo elemento costituzionale, attorno al quale peraltro si è definito l'equilibrio istituzionale di tutti questi decenni? A me pare che i nodi che sono stati posti siano tutti voi scegliete di andare avanti. L'abbiamo detto tante volte anche in Commissione: lo capiamo, ci sono le elezioni europee, vi interessa la propaganda, dovete portare a casa magari qualche voto sull'emendamento per alzare la bandierina; ma davvero non veniteci a dire che questa che state proponendo è una riforma condivisa.

Siete partiti da una proposta che era quella del presidenzialismo; le forze politiche che avete incontrato su quella proposta del presidenzialismo vi hanno detto che non andava bene, perché in questa fase storica non andava bene l'elezione diretta. Cosa avete fatto allora? Avete proposto una ipotesi di riforma, il premierato, che incredibilmente è ancora peggiore del presidenzialismo da cui eravate partiti, perché non prevede nemmeno quei contrappesi democratici che esistono in tutti i Paesi in cui appunto c'è il presidenzialismo. Trovo davvero incredibile che questa scelta, questa forzatura così evidente, venga proposta come una mediazione. È la ragione per cui ho detto che dinanzi a tanta protervia non c'è altra strada che quella che abbiamo scelto noi, che oggi si chiama ostruzionismo parlamentare e domani si chiamerà *referendum* confermativo. È stata fatta la scelta evidente da parte delle forze di maggioranza di non cercare nessun terreno possibile di confronto, anche quando da parte delle opposizioni un terreno di confronto è stato offerto ed era esattamente quello di ragionare attorno alla sfiducia costruttiva, ad elementi che potessero incidere sulla stabilità ma anche sulla rappresentanza; l'altra grande questione di cui sembra davvero che voi non vi occupiate. Non ho sentito una parola, infatti, nemmeno una anche in questa replica, su quelli che sono i grandi nodi della democrazia con la quale ci confrontiamo oggi. Nemmeno una parola sul fatto che mezzo Paese non va più a votare. Ma vi siete accorti che metà del Paese non va a votare nemmeno quando si vota del Presidente della Regione? Oppure non vi siete accorti che c'è un astensionismo gigantesco, che coinvolge ormai mezzo Paese? E voi cosa fate dinanzi a questi nodi democratici così giganteschi, che davvero colpiscono le democrazie contemporanee in un modo così clamoroso? Cercate la strada semplice della scorciatoia. Fareste bene anche a guardare cosa sta accadendo, in questi mesi e in questi anni, anche nei Paesi dove esiste il presidenzialismo, anche con il sistema dei Andate a vedere come si sta lacerando una grande democrazia quale era quella degli Stati Uniti d'America, dove, per l'appunto, gli elettorati dei due diversi candidati pensano: uno, che il candidato dell'altro schieramento

Ma lo capite cosa significa, in una fase storica come questa, con democrazie lacerate, espostissime a rischi di torsione antidemocratica, cosa significa insistere su un tema come quello dell'elezione diretta al tempo della crisi dei partiti e dei corpi intermedi? Ma come fate a non capire che questo è un tema gigantesco? Come si fa a citare Mortati, che parlava del premierato quando esistevano i partiti di massa, che coinvolgevano milioni di persone e che erano loro l'anticorpo e il contrappeso? Ma come si fa a non vedere la differenza gigantesca tra mondi? *(Applausi)*. Basta, ma veramente basta con la propaganda! Basta con la propaganda! Si farebbe meglio a dire: questa è la nostra bandierina ideologica, che ci serve per parlare ai nostri elettori, che dobbiamo motivare ad andare a votare alle elezioni europee; poi, magari, il 10 giugno ne parliamo in un altro modo. Fareste molto più bella figura.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, le ragioni di contrarietà al provvedimento in discussione le ha illustrate nel suo lungo intervento la senatrice Maiorino. Io non aggiungo altro, se non che se non che il non passaggio agli articoli sia anche a tutela di una maggioranza che dice che sta rispettando il proprio programma elettorale. Allora, o adeguate la norma o adeguate il programma, perché dicono due cose molto diverse. Per questi motivi, sosteniamo

La proposta è di non passare all'esame degli articoli, ma, alla fine del suo intervento, egli ha fatto riferimento

***Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica***